finestra"). È stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della salute*: «Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario» finestra"). Un riferimento a quanto accaduto ieri. Credo che con gioia e commozione abbiamo appreso della liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo. A lui, ai suoi familiari e ai suoi colleghi va il nostro abbraccio; a coloro che, nelle diverse posizioni e responsabilità, hanno contribuito alla sua liberazione il nostro convinto ringraziamento; alle forze politiche, nessuna esclusa, che hanno trepidato con noi e hanno manifestato con unità di intenti e di posizioni, che ha grandemente contribuito al positivo esito di una trattativa complessa e difficile, vanno il segno del nostro compiacimento e il nostro ringraziamento. Non posso però non ricordare con dolore che questa drammatica vicenda ha visto un collaboratore afghano di Mastrogiacomo barbaramente ucciso e un altro del quale è al momento incerta la sorte. Fatti, questi, che non possono non addolorarci e rispetto ai quali esprimiamo la commossa solidarietà a coloro che ne sono stati colpiti e alle loro famiglie. Il Senato è alla vigilia di un importante dibattito su un tema, quello della missione in Afghanistan, sul quale le forze politiche avranno modo di misurarsi liberamente. È mio augurio che anche in questa occasione potrà manifestarsi quella forte unità di intenti che, come ho voluto ricordare, è una delle ragioni forti sulla quale si è potuta fondare la liberazione di Daniele Mastrogiacomo. Questa è una nota che il presidente Marini mi ha chiesto di consegnare all'Assemblea.

La sua morte non è rimbalzata sulle prime pagine dei giornali, è rintracciabile soltanto in due o tre righe in tutti i servizi giornalistici, eppure si tratta di un uomo, di un uomo coraggioso. La moglie dell'autista di Mastrogiacomo ha abortito per il dolore. Io qui voglio ricordare anche queste vittime della barbarie e voglio altresì ricordare che per salvare una vita umana si negozia sempre: si negozia per Mastrogiacomo, si è negoziato per Giuliana io sono tra quelli che erano favorevoli al negoziato anche per salvare la vita di Aldo Moro. Signor Presidente, vorrei che il Senato qui, oggi, potesse dare un esempio di solidarietà solidarietà umana verso un uomo che ha dato la sua vita per fare in modo che il mondo sapesse e conoscesse.

comunicazione delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo che, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 aprile 2007. Per quanto riguarda la seduta pomeridiana odierna, è stato anzitutto stabilito che, dopo le mozioni sull'accattonaggio minorile e sugli ufficiali in ferma prefissata, la prevista discussione sulla mozione Polledri ed altri sull'industria conserviera del pomodoro sia ampliata al fine di ricomprendere anche mozioni sull'industria agroalimentare, tra cui quella della senatrice De Petris sull'etichettatura dell'olio d'oliva e del senatore Marcora. Domani mattina resta confermata alle ore 9,30 la chiama per l'elezione di due senatori Segretari, con urne aperte fino alle ore 12,30. È stata invece rinviata ad altra data la votazione per l'elezione dei componenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Dopo la chiama, il Governo riferirà sulla liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo. Potrà successivamente intervenire un oratore per Gruppo per 10 minuti ciascuno (15 minuti al Gruppo Misto). A conclusione di tale dibattito sarà data la parola ai relatori per riferire sul decreto-legge recante rifinanziamento delle missioni internazionali. Sarà quindi aperta la discussione generale che proseguirà nel pomeriggio e, per concludersi, eventualmente anche nella seduta antimeridiana di martedì 27 marzo. A partire dalla seduta pomeridiana dello stesso giorno avranno inizio le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno, che proseguiranno in tale seduta fino al voto finale. La seduta potrà pertanto protrarsi anche oltre il consueto orario. L'ordine del giorno di domani mattina è integrato con lo svolgimento di un'interrogazione urgente sollecitata dai Gruppi. Fermi restando gli argomenti già previsti per la prossima settimana, tempi e modalità di discussione del decreto-legge sulle liberalizzazioni ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - saranno definiti dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Per quanto riguarda la settimana prima di Pasqua, il Senato sarà convocato nel pomeriggio di martedì 3 e nella giornata di mercoledì 4 aprile (giovedì 5 solo se necessario) per l'eventuale esame del decreto-legge sulla violenza negli stadi, ove modificato dalla Camera dei deputati, nonché della mozione Bianconi ed altri sulla medicina di genere e del bilancio interno e rendiconto del Senato.

sono state incarcerate circa quaranta persone che sfruttavano un gruppo di bambini abbastanza vasto. Si trattava di circa 25-27 bambini appartenenti in realtà alla comunità rom, a vario titolo di parentela, sfruttati in maniera massacrante, lasciati sulle strade fino a dodici ore, in condizioni igienico-sanitarie assolutamente insopportabili

noi, cosa possiamo fare? Abbiamo fatto tanto, ma il Governo deve prendere un impegno politico serio: qui parliamo di impegno politico, di volontà politica. Le città si stanno dotando di centri di assistenza attivi 24 ore, in modo che il bambino preso della strada possa essere accompagnato in un centro adatto a lui, dove possa essere verificato il suo stato di salute e la condizione da cui proviene, cioè il luogo di appartenenza, il campo nomadi da cui proviene. Queste sono

ti perdono. È impensabile che sulle strade italiane ci siano ancora donne che fingono di allattare bambini che cambiano continuamente: potrei citarvi un caso di cui sono stata diretta testimone, quello di una donna che si è trovata ad allattare nel giro di un mese bambini di età completamente differente completamente differenti, quindi assolutamente non appartenenti a lei. Di fronte a tutto ciò, che fare, signor Presidente, signori del Governo? Non c'è altra strada che applicare le leggi e rendere lo Stato italiano finalmente degno di questo nome. Esiste la Convenzione di New York, che abbiamo ratificato; esiste la Convenzione dell'OIL contro lo sfruttamento delle peggiori forme di lavoro

aiutare ad accertare la reale presenza della piccola e media criminalità dietro questi bambini. E allora, che cosa vogliamo fare: vogliamo fingere ancora, vogliamo fingere che la questione non ci riguardi? Quando una delle nostre famiglie o uno dei nostri cittadini italiani cerca di capirne di più e telefona al «112» o al «113», gli viene risposto regolarmente: e che ci possiamo fare? Dove li possiamo portare? Anche sulla questione dell'accertamento di maternità o paternità:

si sta discutendo proprio di questo. Allora, vogliamo dotarli di documenti specifici di riconoscimento? Vogliamo fare in modo che non ci siano sempre bambini sottratti, anche bambini italiani? Vogliamo che la storia dei due fratellini siciliani o della bambina di Potenza o del bambino di Milano non si ripetano più? Ebbene, non abbiamo altro sistema che intervenire, visto che anche la Corte di cassazione ci chiama ad un intervento diretto, visto che siamo posti, noi, di fronte alle nostre dirette responsabilità. Signori del Governo, non è pensabile un atteggiamento, per così dire, di estraneità, non è pensabile che ancora una volta cerchiamo di fare finta di niente. La Commissione bicamerale per l'infanzia nella precedente legislatura produsse un atto d'indirizzo

mozione a prima firma della presidente Serafini io mi impegno, come responsabile oltre tutto del mio partito sulle politiche dell'infanzia,

Facciamo qualcosa. Non è possibile che ancora una volta passiamo di fronte alla solita madre con il solito bambino, al solito bambino con l'organetto, al solito bambino che addirittura viene infilato nelle chiese al momento della questua (anche questo mi è capitato di vedere) e che viene regolarmente picchiato

Signor Presidente, lo sfruttamento delle bambine, dei bambini e degli adolescenti è qualcosa che muove molto di più dell'energia necessaria per accurate analisi e ragionevoli proposte per contrastarlo. Lo sfruttamento, quando si applica all'infanzia e all'adolescenza, ha a che fare con una sottrazione doppia. Ogni essere umano ha diritto alla propria integrità fisica e psichica; quando questa è ferita, la persona ne esce sempre diminuita. Ma l'adulto ha la possibilità, la forza di ripristinare la propria interezza, i bambini no, sono veramente senza scampo, la loro forza non è sufficiente. Quando gli adulti che devono provvedere al loro benessere non sono capaci di protezione, o addirittura sono essi stessi coloro che attentano alla loro tutela, allora gli altri, come singoli o come comunità, devono intervenire. L'accattonaggio è una forma di sfruttamento, tra le peggiori. Determina, con le altre forme di sfruttamento più vicine, ad esempio il lavoro minorile, la sottrazione dei bambini a quella che dovrebbe essere la loro vita: il gioco e l'istruzione. Il concetto di infanzia, nei tempi moderni, nasce proprio con la separazione dei bambini dagli adulti, con l'istruzione. La presenza, ancora oggi, del lavoro minorile risulta intollerabile, perché contrasta con l'idea stessa di infanzia come età riconosciuta per la formazione e per lo sviluppo della personalità. La stessa civiltà di una nazione è data proprio dal consentire la salvaguardia di questa età e un Paese è tanto più forte in quanto è in grado di esprimere una politica che non si limiti all'oggi, non rimpicciolisca e non circoscriva l'azione pubblica all'immediato. Alcuni investimenti collettivi hanno un costo immediato, mentre i benefici sono futuri e lontani, distribuiti nell'arco della vita o addirittura di generazioni. C'è bisogno di una politica che guardi lontano; è necessario un lungimirante investimento sul capitale umano: quello più efficace e più in grado di incidere sulla diseguaglianza è quello che parte con i bambini e l'istruzione è leva decisiva per contrastare il peso dell'eredità sociale e affermare le pari opportunità. Per questo il lavoro minorile e la dispersione scolastica vanno combattuti. E con altrettanta forza va combattuto l'accattonaggio, aspetto degradante dell'uso di minori a fini di lucro. A differenza del lavoro minorile, già di per sé fenomeno gravissimo, l'accattonaggio - in tutte le sue forme - è ancora qualcosa di diverso, presuppone una perdita di dignità dei bambini. Il maltrattamento che bambini e adolescenti subiscono è di natura fisica, abbandonati per ore, con ogni tempo, per strada, ma è anche psichica. Non dobbiamo pensare che il disagio dei bambini non sia anche di questa natura. Loro non hanno scelto l'accattonaggio, sono gli adulti che lo hanno scelto per loro, spesso i loro genitori e parenti. Come si possono difendere? Quando si parla di patto tra generazioni, dobbiamo sapere che bisogna includere anche chi non è in grado di stipulare alcun patto. Questo riguarda tutti i bambini e soprattutto quelli che hanno minori possibilità di difendersi. La Convenzione ONU ha chiesto agli Stati di andare oltre i propri confini in relazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cosicché le stesse legislazioni nazionali devono considerare i bambini e gli adolescenti come cittadini a prescindere dal loro Paese di provenienza. L'infanzia impone alla cultura politica di tenere insieme due dimensioni che la vecchia cultura statale aveva trascurato. Queste due dimensioni sono il globale e il locale. La più grande attenzione concreta che si può dare alla cura dell'infanzia in un territorio, Comune, Provincia o Regione, non può essere disgiunta da una cura dell'infanzia che non ha cittadinanza, e viceversa. Proprio per questo i diritti fondamentali hanno trovato, prima di tutto, e spesso in anticipo sulle sensibilità culturali dei diversi Paesi, il loro luogo nella legislazione internazionale. L'infanzia vuole uno sguardo cosmopolita. Obbliga le comunità a guardare oltre lo Stato e quindi oltre i confini stessi della cittadinanza. La Convenzione dell'89 afferma che alcuni diritti fondamentali sono riconosciuti «ad ogni fanciullo che dipende dalla giurisdizione» dello Stato-parte, quindi anche a tutti i bambini e ai ragazzi stranieri presenti nel nostro Paese. Da ciò deriva un divieto di discriminazione sulla base della cittadinanza, principio dichiarato dalla stessa Carta di Nizza. Tutti i diritti di tutti i bambini devono essere quindi fondati sulla base della loro presenza in un Paese, indipendentemente dalla cittadinanza. La tutela della loro integrità, il diritto alla propria famiglia e a vivere nel proprio Paese, il diritto ad essere ospitati e tutelati nei Paesi non di provenienza, condizionano, e devono farlo in modo sempre più adeguato, la legislazione e gli atti dell'insieme dei soggetti pubblici e privati per contrastare l'abbandono, la tratta, ogni tipo di sfruttamento dei bambini e degli adolescenti, a partire dall'accattonaggio. Nelle nostre città il fenomeno dei bambini che esercitano l'accattonaggio e di donne che chiedono l'elemosina con dei bambini in braccio o accanto a loro è reale e visibile. L'accattonaggio interessa, in particolare, soprattutto quei gruppi di zingari profughi nell'ultimo decennio dai tradizionali luoghi di residenza (Kosovo, Romania, eccetera), che sono venuti in alcuni Paesi, fra cui l'Italia. Si sono aggiunte anche altre forme, di ben maggiore gravità, di sfruttamento, in cui adulti stranieri che non sono parenti prendono dalle famiglie di origine dei bambini che utilizzano in Italia per chiedere l'elemosina. In tutti i casi questi bambini subiscono gravi pregiudizi per la salute, per la mancata integrazione con gli altri bambini nell'asilo e nella scuola, per l'impossibilità di costruirsi un loro futuro e, talvolta, per la lontananza dai genitori. I bambini vivono quasi sempre in condizioni di inadeguatezza per gli alloggi nei campi e nelle baracche. Secondo i dati del Ministero dell'interno per gli anni 2003-2005, elaborati dall'Istituto degli innocenti, l'uso di minori in attività di accattonaggio «garantisce rilevanti guadagni alle famiglie dei minori e movimenta enormi introiti per le organizzazioni criminali che lo gestiscono». Le stesse forze di polizia stimano il ricavo medio in 100 euro al giorno per bambino. Ai bambini di origine Rom che vengono costretti ad operare in organizzazioni strettamente familiari si sono aggiunti ormai da anni bambini di origine albanese e rumena che vengono affidati dalle proprie famiglie a vere organizzazioni criminali che si occupano di farli entrare in Italia. Data la sua complessità, il fenomeno è ancora per lo più statisticamente sconosciuto. Tra i dati ad oggi disponibili si hanno quelli che riguardano le segnalazioni alle forze di polizia aggiornate all'anno 2005. Si contano in Italia 455 segnalazioni per impiego di minori in attività di accattonaggio, di queste, 449 riguardano denunce, è necessaria una continua azione per contrastare una concezione, presente spesso nelle comunità di provenienza di molte bambine e bambini, secondo cui l'accattonaggio non è da considerare dannoso per i bambini, bensì un positivo e normale contributo per sostenere economicamente le famiglie;

Per la Cassazione "è evidente che imporre al minore o anche semplicemente consentirgli un sistema di vita non adeguato alle sue esigenze e anzi in contrasto con queste, lasciandolo esposto sistematicamente ai rischi della vita di strada" significa "determinare nella vittima uno stato di sofferenza fisica e morale, avvertito, proprio perché frutto di una condizione abituale e persistente, come intollerabile". Né può evocarsi, conclude la Cassazione, per la concessione delle attenuanti, "l'etica dell'uomo", affermata "sulla base di opzioni sub-culturali relative a ordinamenti diversi dal nostro. Tale riferimento a principi di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia deve cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi di base del nostro ordinamento";

Così come il processo di integrazione europea che si è irrobustito con l'ingresso di nuovi Paesi - alcuni dei quali, come la Romania, sono Paesi di provenienza di un numero non irrilevante di bambini - pone la questione in termini nuovi. Le cose da fare sono molte. Queste secondo la mozione da noi presentata le priorità: disporre un'indagine conoscitiva sul fenomeno; disporre dei piani di sostegno economico e abitativo di integrazione sociale delle famiglie; sensibilizzare, formare e coordinare le forze dell'ordine sull'assoluta necessità di un intervento in tutte quelle situazioni in cui i bambini sono utilizzati da terzi per l'accattonaggio o sono oggetto di tratta; istituire un fondo specifico con risorse aggiuntive e promuovere un coordinamento interistituzionale nazionale che definisca i compiti e gli indirizzi delle diverse articolazioni dello Stato e delle relative amministrazioni; sviluppare rapporti di cooperazione e stipulare accordi specifici con quei Paesi, a partire dalla Romania, che hanno fatto il loro ingresso nella Comunità Europea; verificare l'opportunità dell'istituzione di un apposito numero verde che faciliti una maggiore protezione dei bambini dall'accattonaggio.

La Cassazione, nel testo di cui ho parlato poco fa, fa riferimento al disagio dell'adolescente che ha espressamente fatto richiesta di essere allontanato non solo dallo zio ma dalla stessa città in cui viveva. E' proprio a partire da quel disagio che sono da assumere interamente le parole che Kofi Annan, aprendo la sessione speciale dell'ONU sull'infanzia «Un mondo a misura di bambini», ha detto, rivolgendosi ai bambini e adolescenti e traendo un bilancio delle cose fatte e delle molte che restano da fare: «Avete diritto «Avete diritto a una vita libera dalle minacce della guerra, dell'abuso e dello sfruttamento. Questi diritti sono ovvii. Eppure noi, gli adulti, abbiamo fallito nel garantirvi molti di essi. Uno su tre di voi ha sofferto di malnutrizione prima dei cinque anni. Uno su quattro di voi non è stato vaccinato contro nessuna malattia. Quasi uno su cinque di voi non va a scuola; e tra quelli di voi che vanno a scuola quattro su cinque non riusciranno a completare la quinta classe. molti di voi hanno visto violenze che nessun bambino dovrebbe vedere. Tutti voi vivete sotto le minacce del degrado ambientale». Sono parole durissime, colleghe e colleghi, ma vere. Per questo non dobbiamo avere indulgenza verso chi ritiene morale che si rubi o si neghi l'infanzia. Restituire l'infanzia ai bambini significa restituire loro la possibilità del gioco e dell'istruzione e di vivere il presente con dignità e con la fiducia che gli adulti e la comunità sapranno sapranno proteggerli considerando i loro diritti come il loro bene più prezioso. Signor Presidente, non si può trattare in modo semplicistico un problema complesso, soprattutto non si può pensare di stroncare un fenomeno intollerabile come quello dell'accattonaggio dei bambini e delle bambine, che, proprio perché non può essere da loro scelto e spontaneo, il più delle volte altro non è che una violenza e una riduzione in schiavitù, proprio a partire dalla loro innocenza e dalla loro debolezza. Non si può stroncarlo con la mera repressione di ciò che è visibile, colpendo gli ultimi anelli della catena, quasi sempre i più deboli ed essi stessi vittime di situazioni di sfruttamento. Ma soprattutto non possiamo pensare di intervenire su un problema di questa portata, umana e sociale, senza conoscerlo e provare ad analizzarlo e scomporlo nelle sue parti e nelle diversissime fattispecie che si celano dietro ad ogni bambino che si avvicina tendendo la mano. Non possiamo pensare che ci sia una soluzione taumaturgica ad un fenomeno così vasto e odioso o che un unico attore, sia esso lo Stato o la giustizia, possa risolverlo, tantomeno con la sola repressione, una violenza che si perpetua sotto l'occhio complice di ciascun di noi o peggio con la nostra distratta connivenza. Come ogni mercato, infatti, anche nel mercato dell'accattonaggio dei bambini c'è una domanda e c'è un'offerta (un bambino che «fa manghela» porta a casa mediamente 100 euro al giorno; è una gallina dalle uova d'oro per chi lo sfrutta, sia la sua famiglia, sia, e di questo parlerò più diffusamente dopo, la criminalità internazionale organizzata), ma, come ogni mercato, come quello della prostituzione, come quello della droga, è sostenuto da chi lo paga. Così siamo noi, il più delle volte sostenuti dalle migliori intenzioni, molte volte dalla cattiva coscienza, a rendere redditizio mandare un bambino a chiedere la carità. Se tutti i cittadini, improvvisamente e concordemente, smettessero di dare soldi ai bambini, offrissero loro qualcosa da mangiare (un giochino, un dolcetto, un sorriso o una parola amica), ma per nessun motivo soldi, in poco tempo questo mercato si sgonfierebbe. Certo, non finirebbe lo sfruttamento dei bambini, il malaffare troverebbe immediatamente altre vie per sfruttare i piccoli, magari anche peggiori, ma questa intanto non avrebbe più cittadinanza. accanto a questo, ciascun cittadino o cittadina che incontra una bambina o un bambino intenti ad accattonare dovrebbe rendersi parte diligente sia informandoli del fatto che non è giusto (spesso quei bimbi non lo sanno, spesso nessuno glielo ha mai detto), sia chiedendo loro chi è l'adulto che li ha in carico (aspettiamoci però una risposta bugiarda, perché tutti i bambini così deprivati sono stati costretti a crescere in fretta e a diffidare di tutti), sia avvisando chi di dovere, dal vigile, all'ente locale, ai servizi specifici.

che si lava la faccia con l'acqua fredda, così si sveglia. Credo che la maestra che vede quel bambino assonnato, che non può stare attento alle lezioni se è andato a letto all'una di notte, non si stia facendo parte diligente per farsi carico, come tutti noi dovremmo fare, di ogni bambino. Insomma, nessuno di noi, se pensiamo realmente che l'infanzia sia un bene comune e che il futuro del mondo dipenda anche da noi, dovrebbe mai girare senza avere in tasca una merendina o il numero dei servizi sociali, o, dove c'è, del garante dell'infanzia. questo sia uno dei problemi più grandi del nostro Paese: siamo ancora inadempienti, siamo rimasti l'unico Paese in Europa a non aver istituito la figura nazionale del garante dell'infanzia, cioè una figura che si prenda a cuore specificatamente, ogni volta che i diritti di un bambino sono conculcati. Credo quindi, per questo mi rivolgo alla Presidenza, che siccome ci sono numerose proposte di legge presentate tutti i Gruppi parlamentari su questo tema, sarebbe il caso di metterle in discussione e di arrivare al più presto Dobbiamo però porci anche altri obiettivi; obiettivi politici, ma non per questo meno concreti e concretamente attuabili: prevenire e intervenire contro la tratta, facendolo a partire da un approccio basato sui diritti umani e su quelli dei bambini e delle bambine, ponendo particolare attenzione alla protezione della vittima, attraverso la promozione e la protezione dei diritti di ogni bambino e bambina e della sua dignità. Innanzitutto però, credo che si debba suddividere il fenomeno in due situazioni che, pur dando vita a risultati simili, sono completamente diverse per i problemi che evidenziano. È necessario distinguere i bambini che chiedono l'elemosina insieme alle loro famiglie da quelli che sono vittime della tratta e ridotti in schiavitù. Il bambino non ha libertà e il rispetto dei suoi diritti e della sua libertà va comunque tutelato, ma i problemi e soprattutto le possibili soluzioni sono completamente diversi. Il bambino che mendica con i suoi genitori o da solo spesso fa parte di un nucleo familiare povero, economicamente e socialmente. Non dobbiamo criminalizzare nessuno per questo. Ogni bimbo o bimba nei primi anni di vita sta insieme alla mamma e al papà mentre lavorano e non può essere certo criminalizzato il fatto che per alcuni genitori l'unica fonte di reddito sia l'accattonaggio, ma va, semmai, fatto qualsiasi sforzo per sostenere la ricerca di una fonte di reddito adeguata alle necessità della famiglia e questo, direi, senza falsi moralismi. Ho parlato recentemente con una mamma rom che stava mendicando ad un semaforo con un bambino di cinque mesi attaccato al seno; ne abbiamo parlato molto, abbiamo visto per lei delle soluzioni; i vigili l'hanno avvicinata, le hanno detto più volte che se l'avessero trovata ancora con il bambino attaccato al seno l'avrebbero denunciata, le avrebbero portato via il bambino; insomma, tutta una serie di cose che, all'atto pratico, sono impossibili e sbagliate. Quella donna si è così spaventata che lascia il bambino al campo *rom*, ha smesso l'allattamento, prende il treno ogni mattina, va a chiedere l'elemosina a Padova per non essere riconosciuta,

allora, sia il caso non tanto di criminalizzare o spaventare qualcuno con informazioni più o meno vere, ma di domandarci, per esempio, se il nostro Paese tuteli o meno la maternità per sapere perché quella mamma con un bambino di cinque mesi non goda di alcun sostegno economico o sociale come tutte le altre donne che accedono alla maternità. ancora. Diventa indispensabile l'adozione, come avviene in molti altri Paesi anche europei, del reddito di cittadinanza per i bambini. Se il nucleo familiare in cui un bambino nasce e cresce non è in grado per problemi di ordine sociale, psicologico, ambientale o economico di salvaguardare e garantire tutti i suoi diritti - e non vi è dubbio che la povertà metta in discussione ogni diritto - uno dei compiti della società è sostenere quei bambini e quelle bambine. Molto ci si affanna da destra e, qualche volta, anche da sinistra ideologicamente sulla famiglia, ma poco si fa per concrete politiche di sostegno indirizzate alle persone che nella famiglia sono La cura dei bambini non può continuare ad essere ritenuta un affare privato, lasciata alle soluzioni individuali, all'arrangiarsi delle reti familiari. Ogni bambino rappresenta un valore incommensurabile non solo in sé, non solo per la famiglia in cui si trova a nascere, ma per l'intera società. Insomma, ogni bambino in quanto tale, è un valore sociale che va difeso e sostenuto dall'intera società anche economicamente, se si trova in una situazione di bisogno. Oggi vi è piena consapevolezza - anche se, purtroppo, non altrettanta piena attuazione - dell'importanza di tutelare i diritti dei bambini. L'infanzia è un valore che va tutelato come un bene comune, trovando nuove forme sociali e istituzionali. Questa è una delle nuove sfide che il nostro sistema politico e sociale e il nostro Governo si trova a dover affrontare, se non vuole continuare a basarsi sulla facile scorciatoia di abbandonare i bambini più deboli alla responsabilità esclusiva dei loro genitori. Il benessere dei bambini e delle bambine deve diventare, perciò, il perno delle scelte politiche, particolarmente in ambito sociale ed economico. La Convenzione sui diritti del fanciullo sancisce espressamente per ogni bambino e bambina il diritto alla salute, a vivere liberi da condizioni di povertà e degrado,

La garanzia di una esistenza libera dal bisogno e la conseguente necessità di corrispondere a chi versa in condizioni disagiate un sostegno economico di base rappresenta una delle priorità per tutti gli Stati che sono, quindi, tenuti a garantire che bambini e adolescenti possano godere di un reddito minimo garantito o da parte del nucleo familiare di origine o, se questo non può, con intervento dello Stato, se gli adulti cui sono affidati non possono assicurare la libertà del bisogno. non mi addentro ulteriormente nella materia perché esulerei dall'argomento di oggi, ma sarebbe anche necessario sostenere i genitori e gli altri familiari nella ricerca di un lavoro adatto e sostenibile, inserire i bambini nella rete dei servizi sociali, nei nidi, nelle scuole materne al pari con gli altri bambini italiani. Questo per quanto riguarda i bambini che fanno accattonaggio insieme con le loro famiglie di origine. Di tutt'altro tenore, invece, devono essere le considerazioni quando il bambino sia sfruttato da estranei. leggerò un caso giornalistico (tra i troppi) per capire di cosa parliamo, di quale fattispecie di tratta: «Costringevano tre minorenni, un ragazzino e una ragazzina di tredici anni e una bambina di sette, all'accattonaggio guadagnando ognuno in media 100 euro al giorno. Per loro una vita d'inferno; dormivano in tenda, in mezzo alla strada, ma a volte anche nei locali fatiscenti di una ex fonderia. Come bagno, in caso di necessità, una cabina telefonica. Anche quando le temperature erano rigidissime loro erano lì, negli incroci più trafficati, a chiedere l'elemosina. A sfruttarli erano tre rumeni, tutti regolari, arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di tratta di minori. Sia gli adulti, sia i bambini provenivano da una zona della Romania l'Italia rappresentava soltanto un luogo di passaggio, essendo già stati prima in altre città. Agli agenti i tre fermati hanno dichiarato di essere i genitori e un cugino dei minori, ma la polizia ritiene che non sia così, ad accertarlo sarà l'esame del DNA. I bambini venivano trattati in modo disumano e minacciati se non guadagnavano abbastanza. Ogni mezz'ora, al massimo quaranta minuti, dovevano consegnare le elemosine raccolte. I minori sono stati affidati ad un istituto». Questa la fredda cronaca di uno dei tanti esempi che abbiamo nelle nostre città, eppure in Italia esiste una legge importante a questo proposito, l'abbiamo approvata nella scorsa legislatura, la n. 228 del 2003, «Misure contro la tratta di persone» che devono, a maggior ragione, valere anche per i bambini. Questa legge interviene, almeno sulla carta, su molti versanti, innanzitutto sul versante della prevenzione, perché da al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, il compito di attuare politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi di origine di questi bambini vittime ed anche di organizzare incontri internazionali e campagne di sensibilizzazione. Interviene, questa legge, anche in maniera interessante ed intelligente sul versante della protezione delle vittime, perché vengono previsti programmi d'emergenza per l'assistenza alle vittime, in modo da garantire alloggio, vitto e assistenza sanitaria, ma istituisce pure un Fondo nazionale per le vittime della tratta che dovrebbe essere finanziato con i beni confiscati a conclusione di procedimenti giudiziari, e poi questa legge prevede, sul piano sanzionatorio, oltre alla definizione specifica di tratta di esseri umani, disposizioni specifiche nel caso di abuso a danno di minori, disponendo l'aggravamento delle pene da un terzo alla metà (quindi siamo dai 5 ai 15 anni se il minore sfruttato e trattato è minore di anni 18).

per tratta di minori vi sono state 279 denunce, nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge le denunce sono raddoppiate. A questa legge, si accosta anche una sentenza che ha stabilito che può essere disposto il carcere preventivo per chi sfrutta i minori mandandoli a chiedere l'elemosina. Tale sentenza, quindi, riconosce che costringere i bambini a mendicare, quando a farlo non sono parenti, è riduzione in schiavitù. Ma quello che più conta sono le azioni concrete che in alcune parti del nostro territorio sono state attivate grazie a questa legge e che andrebbero generalizzate ovunque ci sia un bambino. Per esempio, abbiamo avuto l'anno scorso in Commissione infanzia, il Centro per la lotta all'accattonaggio minorile del Comune di Roma: è un centro che è stato istituito con i fondi della legge n. 285 del 1997 (e vorrei ricordare che quella legge non era stata più finanziata dal precedente Governo e ora mi auguro questo Governo vorrà Grazie a questa legge si è aperto il Centro contro l'accattonaggio che ha come finalità quella di togliere immediatamente i minori dalla strada per inserirli in un contesto più accogliente, lontano dallo sfruttamento e dando loro stimoli concreti per il cambiamento delle loro esistenze Nel Centro si prevede un approccio multidisciplinare di intervento, esso viene gestito in collaborazione dalla Polizia municipale, dalle Forze dell'ordine, da un'unità di strada, da un'unità di intervento per le famiglie, dalla rete ospedaliera

A livello locale, sempre a Roma, è stato istituito un centralino telefonico (con il n. 0661532567) proprio contro lo sfruttamento dei minori dediti all'accattonaggio. Sempre nella capitale, si è avviato un lavoro di informazione e prevenzione nei campi rom e nei luoghi di frequentazione ed insediamento di stranieri, effettuato anche grazie alla quotidiana collaborazione con la Polizia municipale e con l'associazionismo. C'è poi il Comune di Torino, tra i primi in Italia ad aver adottato il piano dei servizi sociali di zona, che ha rafforzato lo stretto rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato in raccordo con servizi comunali, ha consentito di avviare un controllo capillare e una capacità d'intervento sui singoli casi e ha permesso anche un consistente numero di attività e progetti finalizzati alla prevenzione dei rischi, al recupero delle situazioni problematiche e all'inserimento sociale dei bambini. Il Comune di Napoli - credo che il collega Tecce ne sappia qualcosa - ha creato e reso operativi vari interventi di sostegno al nucleo familiare e al recupero dei bambini a rischio con il progetto «I Fratelli di Iqbal», destinato ai minori stranieri non accompagnati e presenti sul territorio cittadino. È emersa anche la necessità di interventi localizzati, affidati ai Comuni, finalizzata allo scambio di esperienze e al monitoraggio. Per questo si è creata la «Rete di Comuni», alla quale hanno aderito fino ad ora nel nostro Paese oltre 100 municipalità, prima fra tutte, Napoli.

Ancora, vanno fatti degli interventi di collocamento lavorativo, di collocazione professionale per gli adolescenti e iniziative di sviluppo economico per le comunità e i gruppi di rischio. vanno poi contestualizzati, dando importanza, non solo alle caratteristiche personali dei bambini vittime ed al contesto familiare di appartenenza, ma anche cercando di capire le modalità di reclutamento, di trasporto e l'esperienza di tratta vissuta. Ancora, vanno inseriti dei servizi specifici per i minori vittime in relazione alla loro età, al sesso, alla fase di sviluppo, ai bisogni e alle diverse forme di sfruttamento sofferto. Perché oggi, se ci pensiamo bene, stiamo assistendo ad un'involuzione totale delle condizioni dell'infanzia nel mondo e alla nascita continua di nuove forme di sfruttamento che violano il diritto di ogni bambina a vivere un'infanzia felice e piena. Questo, evidentemente, dipende anche dalla ripartizione sempre più ineguale delle ricchezze mondiali e dalle sacche di miseria - di estrema miseria - che vengono generate, gettando le popolazioni più vulnerabili nelle mani dei trafficanti che godono spesso di un'impunità totale. La nostra mozione prevede alcune cose molto concrete che cerco di riassumere. vuole impegnare il Governo ad attuare dei controlli di identità, di appartenenza familiare accertata e riconosciuta perché alcuni bambini che giungono nel nostro Paese non sono mai stati registrati in nessuna anagrafe: non esistono e, quindi, possono essere oggetto di qualsiasi sfruttamento, fino alla morte. morte. Ricordiamoci che i dati, al 31 dicembre 2005, ci dicono che 1.476 minori stranieri sono scomparsi nel nostro Paese. Ancora, dobbiamo lavorare contro la dispersione scolastica, dobbiamo creare le misure di sostegno ai nuclei familiari di cui ho parlato prima. Dobbiamo altresì intraprendere ed implementare, attraverso gli enti locali, i programmi di prevenzione. Rimando, per mancanza di tempo, alla nostra mozione. Credo che la discussione di oggi sia estremamente importante perché tocchiamo il cuore di un problema che è inaccettabile esista, ma che non può essere risolto con la semplice repressione. *(Applausi dal

Lo faccio con grande convinzione, anche come sottoscrittore della prima mozione, quella che ha come prima firmataria la collega Burani Procaccini. Certamente non lo faccio per consegnare un brandello della mia coscienza a questo dibattito, ma con l'intenzione o la presunzione di contribuire a cercare, non certo una semplice esibizione di pietismo, ma magari la produzione di qualche proposta concreta con la quale affrontare questo complesso problema, talmente complesso che è persino difficile sviscerarlo in quanto investe aspetti umani, sociali, giuridici, politici ed etici. Gli aspetti umani sono quelli che coinvolgono ciascuno di noi quando ogni giorno ci fermiamo ad un semaforo e, con il perentorio cenno del nostro dito indice, neghiamo quella patetica pulitura del parabrezza della nostra vettura, che altro non è che la contropartita di un servizio che nasconde chiaramente il gesto dell'elemosina. In quel momento non neghiamo soltanto un servizio; neghiamo dignità al bambino che ci offre quella prestazione. aspetti sociali, evidentemente se il problema è diventato acuto al punto in cui ci troviamo, i servizi che pure lodevolmente sono stati messi in campo o sono insufficienti o sono inefficienti. In questo senso è l'ente pubblico che deve interrogarsi.

agli aspetti politici, chiediamoci se davvero la politica ha prodotto tutti gli strumenti, tutto quello che può e che poteva mettere in campo per affrontare questo problema su un piano legislativo.

Non ci rendiamo conto che stiamo analizzando non soltanto un caso che induce a pietà o che fa discutere su un piano di carattere giuridico, ma un problema che pone in dubbio e minaccia la dignità di persona di questi bambini nell'età più fragile e decisiva per la loro educazione e per il loro futuro di cittadini; è sulla dignità che l'etica deve intervenire. Allora, quali misure porre in campo? Bisogna intervenire la prima, la più importante, è l'assistenza alle vittime, che sono gli stessi bambini; la seconda è la prevenzione, la vigilanza. Diciamo la verità: molto spesso ci chiediamo come facciano quei vigili urbani, quei poliziotti o quei carabinieri a rimanere indifferenti o a chiudere gli occhi - come si usa dire - di fronte allo sciame di bambini che chiedono l'elemosina o che fanno accattonaggio all'angolo della strada. Chiaramente, anche le forze dell'ordine, al di là di una partecipazione emotiva al problema, sono consapevoli dell'inadeguatezza degli strumenti di cui dispongono. La terza misura va nella direzione della repressione, che non va fatta, colleghi, nei confronti delle famiglie che mettono sulla strada questi bambini, ma delle organizzazioni internazionali che fanno da regìa, non tanto occulta, a questo reticolato indegno, a questa strumentalizzazione. Gli strumenti ci sono: la Carta dei diritti fondamentali di Nizza, la Carta dei diritti del bambino di Treviso, la Carta dei diritti dell'uomo, la Convenzione di New York. Insomma, non possiamo nasconderci dietro il dito di non avere dei riferimenti giuridici. I riferimenti ci sono; occorre ancorare ad essi una coerente convinzione, una determinazione a porli in atto e soprattutto, al di là delle dichiarazioni formali, della partecipazione emotiva, produrre qualche misura che concretamente colpisca all'origine un problema così complesso. Signor Presidente, colleghi, penso che la riflessione di oggi sul drammatico tema dell'accattonaggio minorile, dei soprusi che i bambini sono costretti a subire, possa essere un momento alto della vita parlamentare. Noi, tutto il Parlamento, non ci arrendiamo, non ci dobbiamo arrendere all'idea che un bambino o una bambina possano essere costretti ai bordi delle strade a chiedere l'elemosina; quindi, spero che questo sia un intento comune. Proprio la delicatezza del tema richiede uno spirito laico e una grande consapevolezza non solo delle soluzioni possibili, ma anche dei motivi che oggi ci portano a questa discussione. Quello che non sarebbe sopportabile, invece, sarebbero le squallide semplificazioni lombrosiane, quel sociologismo d'accatto che imputa a particolari culture ed etnie una mai dimostrata propensione alla criminalità e all'ingiustizia. Se scadessimo in questa discussione sul filo di un inaccettabile razzismo, non faremmo un buono servizio né a noi stessi, né ai bambini che vogliamo preservare. Bisogna guardarsi in faccia e avere la consapevolezza che questa piaga è l'effetto di processi vasti sui quali dobbiamo intervenire con forza. Il primo punto è l'Europa che è oggi a due velocità, dove si uniscono luoghi di benessere e luoghi di profondo disagio e di intollerabile ingiustizia. Sarebbe troppo facile vedere solo i bambini migranti, siano essi rom o altro, senza pensare al grado di disperazione che questi bambini vivono nei Paesi dai quali fuggono. Se non saremo in grado di prosciugare quella povertà lontana, qualunque intervento repressivo sarà fiacco e di cortissimo respiro. Nel nostro dibattito non possiamo dimenticare quello squarcio nella coscienza europea che è stata la guerra nella ex Jugoslavia. Quei capi *clan* che sfruttano i bambini e quei genitori che li affittano, figure orrende, un tempo avevano un Paese e un lavoro. In Jugoslavia, il fenomeno dell'accattonaggio minorile era marginale, se non inesistente; allora, chiediamoci perché oggi assistiamo a così turpi comportamenti, agli effetti nefasti della guerra, all'idea della violenza come unica leva d'identità. Non abbiamo fatto abbastanza per sanare quella ferita e l'infezione non rispetta i confini. Non si tratta di parlare d'altro, ma di avere la consapevolezza che le ingiustizie portano con sé ingiustizie più profonde e che se non sapremo dare una risposta a queste povertà e a queste disperazioni, dovremo ancora fare i conti con gli effetti della miseria. Nessuno creda di poter scegliere la scorciatoia dell'arroccamento e della chiusura a riccio delle frontiere. L'Europa si fonda sulla libera circolazione di merci, capitali e uomini e già abbiamo ferito profondamente l'impalcatura comunitaria prevedendo uno slittamento, in occasione dell'ingresso dei nuovi Paesi membri, della libertà di spostamento delle persone. Non possiamo immaginare che la povertà sia accettabile solo se è lontana dai nostri occhi, che le nostre aziende possano pagare a Timisoara i lavoratori un decimo di quanto vengono pagati i lavoratori nel nostro Paese purché siano rinchiusi in Stati ghetto. Se qualcuno lo credo, proponga allora che il nostro Paese esca dall'Unione Europea perché questa sarebbe l'unica strada. Serve la repressione, ma serve soprattutto un'incisiva azione sociale. È dimostrato come le dinamiche di oppressione che si costruiscono nelle comunità chiuse (siano esse un campo nomadi, dove gli adulti fruttano i bambini, o la comunità islamica, dove è socialmente accettato picchiare la moglie) siano avviate dalla debolezza dei servizi sociali, da un contesto non accogliente, da un intervento inadeguato di sostegno e come gli aspetti deteriori di queste comunità non resistano di fronte al dispiegarsi di serie politiche sociali. Non è vero che c'è una sola comunità rom che preferisca il campo nomadi ad una casa e a un tetto sopra la testa. Il punto è che oggi le politiche di edilizia pubblica sono ancora troppo deboli ed inadeguate; così come inadeguate sono le politiche volte a disperdere i ghetti che sono una realtà inaccettabile per il nostro Paese, ma sempre più presente. Dai campi nomadi e da interi quartieri acquisiti da alcune comunità, assistiamo al crescere di luoghi dove vivono regole diverse da quelle dell'ordinamento e da quelle della legge, ma solo una seria possibilità di futuro per le figure emarginate consente oggi di spezzare le regole del ghetto. Serve, inoltre, ribadire con forza il ruolo della scuola. Nelle mozioni in discussione vedo solo un breve cenno e ciò mi sembra una sottovalutazione. Noi possiamo affrontare il tema della convivenza delle culture in tanti modi diversi; possiamo pensare che le altre culture si debbano adeguare non solo alle nostre leggi, com'è ovvio, ma anche alle nostre abitudini e ai nostri costumi, oppure possiamo pensare di giustapporre nuove culture alla nostra creando nuovi ghetti. Sarebbero entrambe soluzioni foriere di conflitti e inadeguate alla situazione che il nostro Paese sta vivendo. L'unica opportunità è data dal rispetto delle regole e da una sana apertura al confronto. C'è un luogo dove questo può avvenire: la scuola. Una seria politica contro la dispersione scolastica è il primo intervento contro lo sfruttamento dei minori. L'Italia ha un primato che ci inorgoglisce e che riguarda gli insegnanti di sostegno. Questi garantiscono supporto a tutte le situazioni di difficoltà, anche alle provenienze culturali diverse, ma è necessario che quei bambini a scuola ci arrivino, anche facendo intervenire - dove serve - le forze dell'ordine. Noi abbiamo gli strumenti per debellare questa piaga ma saremo efficaci solo se avremo il coraggio di un intervento a largo spettro: politiche sociali ed abitative per eliminare i ghetti, politiche europee per una maggior coesione sociale nel Continente, politiche scolastiche per riaffermare che la scuola non è solo un'opportunità, ma anche un obbligo, politiche di repressione per colpire gli sfruttatori. Solo se le diverse istituzioni sapranno coordinare gli interventi per un fine comune potremo essere efficaci, ed è l'efficacia che ci chiedono quei bambini di cui oggi stiamo parlando. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, ringrazio sinceramente la senatrice Maria Burani Procaccini e gli amici del suo Gruppo per la mozione n. 60, che ha ad oggetto il fenomeno dell'accattonaggio minorile. Condivido appieno l'iniziativa e chiedo di poter aggiungere la mia firma a quella dei colleghi che l'hanno già sottoscritta. Condivido la vostra mozione perché è senza retorica, ma, in modo puntuale e asciutto, ci richiama ad una realtà che non ha bisogno di essere giudicata e valutata. La realtà dell'accattonaggio dei bambini e degli adolescenti va semplicemente combattuta, e, dove possibile, estirpata alla radice. L'obiettivo della mozione è certamente quello di verificare lo stato delle cose a questo riguardo e richiamare tutti gli apparati e gli organi amministrativi dello Stato e delle autonomie a compiere fino in fondo il proprio dovere. Mi voglio soffermare su alcuni aspetti del fenomeno prima di fare anch'io alcune proposte. L'accattonaggio è parte integrante di alcune culture di popoli nomadi europei, oggi forse soltanto di quelli di religione islamica. È un fenomeno, questo, al quale siamo abituati da sempre, sia nei piccoli centri di Provincia come nelle grandi città, un fenomeno che era entrato a far parte del costume sociale delle nostre città, guardato con sospetto ma mai demonizzato, contenuto nel numero e per certi aspetti tollerato, come fosse quasi un elemento pittoresco della nostra società. Abbiamo sempre assistito all'accattonaggio anche di persone adulte, italiani ed italiane, poveri, malati, che ricevevano così un pubblico e diretto sostentamento da parte della loro comunità di appartenenza. Ma questo quadro quasi romantico è stato profondamente sconvolto negli ultimi decenni. Per prima cosa, il fenomeno si è allargato nel numero dei soggetti, e nella vastità delle manifestazioni, spesso incrociando altre modalità malavitose di piccole criminalità, secondariamente, sono cambiati i riferimenti etnici e sociali. Non sono più gli zingari, anzi questi rappresentano una piccola parte del tutto, ma sono cittadini di svariati Paesi dell'Est europeo, in prevalenza rumeni, che organizzano e gestiscono questa attività. È arrivato il tempo, quindi, di cambiare strategia ed atteggiamento mentale verso l'accattonaggio, in particolare verso quello minorile. Il principio da affermare è che non può più essere tollerato in nessuna forma. Pertanto, la prima azione da intraprendere è di ordine repressivo, per lo meno per contenere il fenomeno ed esercitare quella funzione dissuasiva verso chiunque intenda avviare all'accattonaggio nuovi minori. Esiste una legge in proposito che è già stata opportunamente richiamata: «Misure contro la tratta di persone», la n. 228 dell'agosto 2003, quindi neanche recentissima. La norma all'articolo 1 è lapidaria riguardo all'accattonaggio, prevedendo, se i soggetti coinvolti sono minori, pene che vanno da un minimo di otto-dodici anni ad un massimo di venti-trent'anni, pene pesanti, paragonabili a quelle previste per l'omicidio. Ci stiamo chiedendo quale sia lo stato di applicazione di questa norma e quanti sfruttatori di bambini, costretti a mendicare, abbiano pagato. Essendo l'accattonaggio un'attività necessariamente pubblica, non dovrebbe risultare difficile scoprire un numero considerevole di adulti responsabili, tale da essere questa un'azione efficace, per un adeguato deterrente. Se questa mozione sarà approvata a larghissima maggioranza dall'Assemblea del Senato, o forse all'unanimità, il Governo avrà uno stimolo in più per programmare un'azione forte su tutto il territorio nazionale. Potremmo immaginare una sorta di ampia collaborazione di polizia statale e comunale per assestare un duro colpo al fenomeno e riuscire a scoraggiarlo per alcuni anni almeno. Una costante vigilanza dovrebbe poi prevenirne l'insorgenza. Saremmo però miopi se non analizzassimo il fenomeno anche sul versante sociale e familiare, al fine di offrire soluzioni adeguate e durature nel tempo. Che cosa accadrebbe infatti a un minore se i propri genitori fossero arrestati per averlo messo in strada? Certamente un altro parente o conoscente della sua famiglia o del suo clan, o un qualsiasi losco individuo, sarebbe pronto a prenderlo sotto la propria protezione per continuare a sfruttarlo. Vanno adottati comportamenti e provvedimenti amministrativi e sociali capaci di sterilizzare il fenomeno dell'accattonaggio. Sembrerebbe ovvio, ma sarebbe sufficiente che nessuno facesse più offerte di denaro a chi tende la mano per strada.

Certamente, però, restano i poveri, che invece possono e debbono essere aiutati, attraverso centri adeguati promossi dalla generosità delle chiese, delle associazioni *no profit* e di privati cittadini; su questi, come sempre, vigilano le istituzioni pubbliche. Non aboliremo gli aiuti alla povertà; semplicemente si sposterebbe l'indirizzo da cui può venire un aiuto sottraendolo alla possibilità dello sfruttamento dei minorenni. Questo tipo di modalità è la norma nei Paesi del Nord Europa e anche di tante città italiane. Si tratta solo di crederci e di attuarlo tutti: polizie da una parte, realtà di assistenza e soccorso sociale per i poveri dall'altra. Nei comportamenti sociali da attuare vi è poi anche quello di non farsi prendere dalla facile pietà quando vediamo un bimbo coinvolto nell'accattonaggio, magari in braccio alla madre. C'è quindi un problema di natura sociale che si deve tentare di rimuovere. Per quanto dobbiamo essere rigidi, categorici e determinati nell'applicazione autentica del codice penale, certamente non possiamo non immaginare soluzioni altrettanto determinate quando si tratta di affrontare in positivo progetti volti all'eliminazione del fenomeno, ai problemi di natura culturale e a quelli legati alla naturale inclinazione egoistica, che porta più facilmente a sfruttare i più deboli piuttosto che andare a lavorare per mantenersi. argomenti sono di natura squisitamente soggettivi, ma non possiamo nascondere le difficoltà oggettive che certa immigrazione incontra nell'inserimento socio-economico nella nostra società. pertanto che al massimo di rigore richiesto nella repressione del reato di sfruttamento dell'accattonaggio minorile debba corrispondere un grande impegno nella prevenzione e nell'eliminazione, ove possibile, delle cause che lo generano. Per cominciare, è necessario rafforzare i controlli in entrata nel nostro Paese. Se arrivano famiglie senza un lavoro con bambini o, peggio, minori senza la loro famiglia, è evidente che qualcosa non funziona nella politica e nell'amministrazione deputata all'immigrazione. secondo elemento è certamente legato all'abitazione. So di toccare un argomento immenso, ma se è vero che un numero considerevole di extracomunitari ha acquistato e acquisterà una casa in Italia, si può pensare che l'integrazione funzioni e che forse solo una piccola percentuale di stranieri ha bisogno di un'abitazione, magari assegnata in forme fortemente agevolate. La casa non va data gratuitamente e non va data a gente che non lavora, ma bisogna pensare seriamente a questo elemento per limitare il nomadismo e la precarietà di vita ai quali, normalmente, è legato l'accattonaggio. terzo elemento riguarda i bambini, i ragazzi e la scuola. Essi vanno tolti dalla strada per essere portati a scuola. Anche questa è un'ovvietà, ma ciò va fatto con energia. Cito un'interessante esperienza compiuta a Torino e in altre città italiane quando, durante l'inverno, i bambini di strada vengono fatti vivere in appositi centri predisposti dalla Croce Rossa e dalla Protezione civile, per proteggerli dal freddo delle strade e delle loro stesse *roulotte*, dove a volte per riscaldarsi si finisce per causare gravi tragedie che portano alla morte di intere famiglie. Esiste anche il problema dell'accoglienza a scuola. Bambini e ragazzi di strada non sono normali minorenni extracomunitari: hanno bisogno di un trattamento particolare fatto più di affetto e calore umano che di procedure didattico-scientifiche. C'è da tenerne conto. C'è anche da considerare la questione del lavoro. Forse, piccole e limitate licenze di commercio ambulante per prodotti di merceria o di artigianato locale tipico, per esempio, rappresentare una valida alternativa per chi non è abituato a lavori ad orario e svolti in ambienti al chiuso. Può, questa modalità, Può, questa modalità, rappresentare un passo importante verso la stabilizzazione del lavoro, certamente un passo verso la legalità, molto significativo rispetto alla criminalità ed allo sfruttamento dei minori. allo sfruttamento dei minori. Da ultimo, credo che vada dato un più significativo supporto alle realtà *no profit* che operano a favore dei bambini di strada, degli zingari, delle famiglie nomadi in genere. Non abbiamo alternative. Né lo Stato né i Comuni potranno mai pensare di svolgere un'adeguata azione educativa a favore di queste comunità o di questo tipo di immigrati. Troppo intensa e troppo dispendiosa sarebbe qualsiasi forma di intervento pubblico; lo dico anche in forza della mia esperienza di amministratore locale delegato all'immigrazione: l'attività educativa non può essere svolta in strutture pubbliche. Ringraziamo coloro che hanno deciso di spendere la loro vita a beneficio di queste particolari e difficili realtà; facciamo però la nostra parte come Stato e assegniamo fondi più consistenti allo scopo. La legge n. 228 del 2003 destina due milioni e mezzo di euro a questo fine: mi sembra veramente poco. Possiamo fare molto di più all'indirizzo di coloro che nel tempo hanno dimostrato capacità ed impegno serio a favore dei più piccoli, sfruttati o abbandonati dai loro stessi genitori*.

sarebbero circa 20.000, di cui 8.000 solo nel Lazio, i bambini che chiedono l'elemosina per le strade delle nostre Città. In realtà il dato non è certo e di difficile comparazione: non esistono infatti uffici pubblici né del volontariato sociale in grado di quantificare in maniera certa il fenomeno nel nostro Paese. Una cosa è invece certa: sono quasi tutti immigrati stranieri e tra questi spicca la nazionalità rumena o slava. Molti dei piccoli mendicanti sono mandati a elemosinare da comunità *rom* o da vere e proprie organizzazioni criminali pronte a dare pene esemplari nel caso di un ritorno a mani vuote dopo una giornata in strada. Un giro di affari colossale, che vede coinvolti bambini di tutte le età, dai piccoli addormentati in braccio alla ragazza che pulisce i vetri al semaforo fino ai portatori di *handicap* ed ai gruppi addestrati ai borseggi. Il fenomeno si intensifica nelle grandi città e anche se la mendicità non è più considerato un atto illecito quando tocca i bambini diventa illegale e dolorosamente inaccettabile dal punto di vista morale e sociale, come diverse sentenze hanno sancito nel tempo. Sono proprio queste sentenze a darci la misura e la cifra dello sfruttamento e della soggezione psichica e fisica dolorosamente applicata su questi minori. È stato chiarito dalla Suprema corte che la finalità di sfruttamento di cui all'articolo 600 del codice penale distingue il reato di riduzione a schiavitù e sfruttamento per accattonaggio di minori da altre forme illegali di inibizione della libertà personale; e non è esclusa, come qualche imputato aveva cercato di dimostrare, quando una parte degli introiti dell'accattonaggio vada a beneficio dei bambini offesi dal reato. Spesso questi sfruttatori sono proprio i genitori. La Corte ha anche deciso che il semplice abbandono dei figli a chiedere l'elemosina sul marciapiede da parte di una zingara configura un reato, vista la consapevolezza della madre da una parte e la precocità dei figli dall'altra. I bambini mendicanti sui marciapiedi, oltre allo sfruttamento, devono subire maltrattamenti. Inoltre, non vanno a scuola, non giocano, dormono dove capita, vivono ai margini tra denutrizione e malattie. Ecco perché la mera applicazione del codice penale, cioè una esclusiva azione repressiva, non può bastare. Occorre viceversa un'attività preventiva che punti all'integrazione ma ancora prima al controllo dei flussi migratori. Purtroppo dobbiamo constatare che il baby-accattonaggio, secondo il più recente rapporto fornito dal Ministero dell'interno, si riferisce a comunità rom o marocchine ed albanesi, più legata quest'ultima alla criminalità organizzata che alle pratiche di sopravvivenza familiare degli zingari. Sono recentemente entrata in netta polemica con il sindaco di Roma Veltroni, che, dopo avere sgomberato 28 campi nomadi, ha cercato, con l'aiuto del presidente della Regione Lazio e del Ministero dell'interno, di dislocare altrove i nomadi e ciò che portano con sé. Abbiamo assistito nel Lazio ad un'autentica sollevazione popolare. Hanno reagito popolazioni fiere della tranquillità e della serenità dei luoghi che abitano, che costituiscono l'unica loro ricchezza. Non dobbiamo meravigliarci, questo atteggiamento di paura e di diffidenza è la logica conseguenza della incapacità dello Stato e degli enti locali a far fronte alla complessità del fenomeno. Sono convinta che occorra praticare al massimo la solidarietà, ma questo assunto porta con sé che non si possa e debba applicare mai la tolleranza nei confronti degli sfruttatori. All'indifferenza di chi passa e preferisce per comodità allungare una moneta, piuttosto che chiamare le forze dell'ordine, non può corrispondere l'indifferenza delle istituzioni. Ecco perché al Ministro e al Governo chiediamo l'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York e della legge n. 228 del 2003, che - tra le misure contro la tratta di persone - prevede esplicitamente il reato di mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola all'accattonaggio, come ha bene evidenziato la mozione n. 60 della senatrice Burani Procaccini, alla quale chiedo di aggiungere la mia firma. Sappiamo però che non è l'assenza di norme il problema, bensì quello della loro applicazione sul territorio con mezzi e risorse. Occorre un adeguato coordinamento delle forze dell'ordine con le forze di polizia locale, il potenziamento degli uffici minori della Polizia di Stato, che possano fungere da pronto soccorso alla delinquenza minorile sia per i reati commessi dai minori, che in pregiudizio dei minori. È poi necessaria una maggiore capillarità nel controllo del territorio, con la presenza fisica e a piedi di agenti, quali ad esempio i poliziotti di quartiere. I servizi sociali dei Comuni devono essere messi in condizione di operare a favore di questi minori, puntando alla loro scolarizzazione, ma ancora prima alla loro salute. In realtà, dopo la soppressione della norma dell'articolo 670 del codice penale, con la legge n. 205 del 1999, l'impiego dei minori ha rilievo penale solo per l'articolo 671: oggi in Italia mendicare con un bambino in braccio non è reato, mentre lo è far mendicare un bambino. Alleanza Nazionale, primo firmatario il senatore Valditara, ha presentato una proposta di modifica del codice penale per reintrodurre il reato di mendicità molesta, ma forse si potrebbero anche inasprire le pene per i reati che riguardano i minori. Al silenzio impotente dei piccoli accattoni, si unisce quello dei tanti bambini violentati fisicamente e non, fuori e dentro le famiglie, dei bambini delle *baby gang*, della criminalità organizzata italiana, dei bambini violati dalla pedopornografia dilagante, di quelli utilizzati anche in Italia come corrieri della droga o come lavoratori sottopagati, o anche semplicemente oggetto del bullismo dei compagni a scuola. È un'infanzia violata anche dalla violenza informativa dei *mass media* e dai ritmi di città che purtroppo non sono più a misura di bambino. Nel vedere un bambino che mendica, non possiamo esimerci dal pensare alla famiglia che forse non ha mai avuto, o che lo sfrutta. Qui è lo snodo della nostra azione istituzionale, questo è il senso del nostro impegno e dell'azione politica. Senza un padre ed una madre responsabili, nessun bambino potrà avere, come è scritto nella Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'UNICEF, quel clima di «felicità, amore e comprensione che sviluppano armoniosamente la sua personalità» e - aggiungo lo renderanno un uomo integro, onesto e civile. Dobbiamo reprimere, quindi, ogni espressione criminale, ma più ancora educare e colmare le distanze culturali e sociali con quelle comunità che, avendo scelto il nostro Paese per vivere, dovranno accettare e garantire l'intangibilità di alcuni diritti, *in primis* quelli dei loro figli, quale irrinunciabile premessa ad un reale processo di integrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho molto da aggiungere rispetto a quello che ha detto molto bene, poco fa, la senatrice Allegrini. Voglio soltanto puntualizzare qualche passaggio. Credo che il futuro dei bambini sia il futuro della nostra società. Negli occhi di un bambino, però, vorrei vedere sempre la gioia di vivere. di vivere. In questo dibattito, invece, è emerso come vi sia una vera e propria industria del crimine ai danni del bambino. Abbiamo sentito parlare di sequestri e di rapimenti per avviare i bambini alla prostituzione.

dell'organo. Abbiamo sentito parlare di un fenomeno agghiacciante, quello della pedofilia. Abbiamo sentito parlare di uno sfruttamento, l'avviamento alla mendacità, che fa del bambino uno strumento per l'arricchimento di queste cosche criminali.

Ci sono già alcune leggi. Penso, per esempio, a quelle che combattono l'evasione scolastica. Facciamole rispettare! Il ministro Moratti, nella scorsa legislatura, qualcosa aveva cercato di fare in questa direzione. direzione. Due sono i concetti forti per sottrarre i minori da questa situazione, l'educazione e la repressione, perché ci vuole anche quest'ultima.

violata? Penso che nei confronti di tutti questi episodi ci debba essere da parte del Governo una reazione molto forte. Vorrei vedere, da domani, perseguiti

oggi parliamo del futuro delle nostre generazioni, di quell'infanzia negata in Italia e nel mondo, che purtroppo vede milioni di bambini sfruttati in maniera veramente vergognosa.

Ma parliamo anche dei bambini di fogna, dei bambini della Romania. Senatore Valditara, speriamo che i nostri colleghi in Europa, quando hanno

L'accattonaggio è una nuova schiavitù, è la schiavitù moderna ed è l'esperienza di oltre 20.000 bambini, questi sono più o meno i dati che si riferiscono all'Italia; per lo più sono stranieri sfruttati, costretti dai *racket*, ma, spesso e volentieri (troppo spesso e troppo volentieri), proprio dai loro genitori. Se non fosse una provocazione eccessiva, bisognerebbe togliere la patria potestà Secondo l'ultimo rapporto del Segretario generale dell'ONU, presentato anche Roma, all'UNICEF e all'Organizzazione mondiale della sanità, la violenza sui minori è un fenomeno che accomuna tutti i Paesi del mondo.

Almeno 50.000 minori sono stati uccisi nel 2002; 223.000 sono stati costretti a rapporti sessuali o comunque a contatti fisici forzati; 218 milioni di bambini sono lavoratori, di cui 126 milioni coinvolti in attività rischiose; 1,8 milioni sono vittime della prostituzione e della pornografia; 1,2 milioni risultano essere vittime del traffico di esseri umani. Non dimentichiamo poi 140 milioni di ragazze che hanno subito mutilazioni genitali.

si fidano e comprende la violenza fisica e psicologica, la discriminazione, il maltrattamento, addirittura la malnutrizione.

in cui i minori vengono impiegati e diventa un profitto per quei personaggi che ruotano attorno a loro. Più o meno, lo dicevano anche i colleghi, un bambino riesce a raccogliere 100 euro al giorno. Quindi, tanti bambini riescono a fare veramente una quantità di denaro incredibile, esentasse e senza grande fatica, anche perché, come dicevo prima, in forma un po' moralistica quando si incontra uno di questi bambini come si fa a non dargli una moneta?

In Italia l'accattonaggio è un fenomeno che è emerso nella metà degli anni Ottanta e ha coinvolto piccoli nomadi; normalmente sono i rom ma provengono anche dall'Est europeo, cui oggi si aggiungono anche i bambini provenienti dal Marocco. Oltre all'accattonaggio, questi bambini sono obbligati anche ad altre piccole attività criminose, quali i furti e lo spaccio di stupefacenti. Vivono per strada in qualsiasi situazione meteorologica, non interessa se poi si prendono l'influenza o il comune raffreddore. Vivono per strada in uno stato di malnutrizione, soggetti a percosse se non guadagnano quanto imposto e quanto previsto da coloro che li hanno mandati per le strade. Rimangono privi di istruzione. Di fatto, sono veramente ridotti in schiavitù. Questi bambini, che sono estremamente redditizi, vengono fomentati da tutto quel fenomeno dell'immigrazione clandestina che anche nel nostro Paese è molto presente. A livello europeo rilevanti sono stati gli interventi normativi contro il fenomeno più ampio del traffico di esseri umani, e in Italia, così come ricordato dalle colleghe, la legge n. 228 del 2003, con le misure contro la tratta delle persone, ha in effetti modificato il codice penale. Con queste norme si punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Anche oggi è stata ricordata l'attenzione che la Corte suprema

spesso la repressione contro questi sfruttatori non è sempre molto adeguata, in primo luogo, perché i piccoli mendicanti vivono in un clima di omertà e di paura che rende difficile capire dove sono allocati, a chi sono affidati e quali maltrattamenti subiscono.

le colleghe hanno rivolto al Governo richieste estremamente ragionevoli; certo, sono complesse e difficili. Immagino che per voi

anche esemplificative di che cosa secondo noi significa, invece, adottare l'infanzia come uno dei beni primari della nostra società. Mancano certamente, o servono certamente, centri di lotta all'accattonaggio nelle diverse città; in alcune città esistono e danno i loro frutti, ma la rete deve essere molto implementata. Serve un miglior approccio multidisciplinare degli interventi

qualsiasi altra azione pensata ed attuata per togliere dalla strada questi bambini è benfatta e rappresenta una grande benedizione. Signor Presidente,concludo il mio intervento ricordando che un bambino nato in schiavitù, che ha vissuto tutta l'infanzia e l'adolescenza in queste condizioni, quando sarà adulto cercherà di esercitare sui più piccoli la stessa violenza subita. Molto è stato fatto, soprattutto negli ultimi anni a livello di diritto internazionale, ma solo la cooperazione concreta e continua tra i vari Stati, solo interventi più incisivi non solo repressivi, ma soprattutto preventivi ed educativi, potranno permettere nel futuro di abbattere definitivamente ogni forma di crimine che abbia come sua vittima principale il bambino. Tutto ciò va fatto per rispettare il pieno diritto all'infanzia; infatti, nessun Paese può definirsi veramente civile se non pone la totale e piena attuazione ed attenzione alla tutela dei bambini, quali beni primari della nostra società.

le leggi dei Parlamenti abbiano dovuto recepire ed applicare i princìpi in essa contenuti. Per lo più, sono stati demandati alle Regioni gli atti pratici, le attività amministrative, i sussidi e gli ausili da offrire ai minori.

Pertanto, anche se risultano dei ragazzoni corpulenti di età indefinibile, fino a prova contraria, tutti questi ragazzi sono minori. Quelle che noi profondiamo nei confronti di questi ragazzi le possiamo definire delle azioni umanitarie? Sicuramente sì, se andassero a buon fine, cioè se si aiutassero dei ragazzi bisognosi, dei bravi ragazzi che si trovano in oggettive difficoltà.

capire e approfittare delle pieghe di questo Stato italiano così attento, che si preoccupa in modo molto preciso di offrire ad ogni minore presente sul territorio tutto quello che dovrebbe offrire una normale famiglia. Cosa abbiamo come ritorno, o meglio, quali comportamenti chiediamo a questi ragazzi?

di un'altra categoria - la consideriamo un'altra categoria - sono ragazzi provenienti per lo più dalle sponde dell'Adriatico, che arrivano a Brindisi la mattina e che la sera sono già nei centri di accoglienza del Nord Italia.

perché non facciamo rispettare la legge italiana che vale per tutte le famiglie, anche per quei genitori - per lo più stranieri - di questi ragazzi che, se fossero genitori italiani, sarebbero finiti già tutti in carcere? Lascio questo quesito aperto, sottolineando, nel

sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio tutti, in particolare, per queste tre mozioni che ci danno l'occasione di affrontare e di ragionare con voi di un tema che al Governo, attraverso i Ministeri competenti, sta molto a cuore. A tale riguardo, abbiamo già avviato alcune azioni, convinti della necessità di far fronte ad un'emergenza che diventa di giorno in giorno più importante e per la quale occorre un'azione coordinata di tutti i Ministeri, ma anche un'azione coordinata con gli enti locali - come è già stato ricordato - e con le associazioni che di questi temi si occupano. Come ricordato nelle differenti mozioni, l'Italia, per contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei minori, si è dotata di un articolato sistema di misure per la repressione dei reati, quali la riduzione in schiavitù, la prostituzione, la pornografia minorile, il turismo sessuale, la violenza sessuale e gli atti sessuali contro i minorenni. In particolare, per quanto concerne il fenomeno della mendicità infantile, nuove importanti misure, che si aggiungono al quadro legislativo di protezione di minori sono quelle della citata legge n. 228 che ha il fine di combattere, in particolare, lo sfruttamento di minori in pratiche di accattonaggio. Si ricorda, inoltre, che in attuazione del disposto dell'articolo 18, Testo unico n. 286 del 1998, è stato attivato un Numero verde nazionale anti tratta, oggi finanziato dal Ministero per le pari opportunità. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e si compone di una postazione nazionale e di 14 postazioni locali; locali; riceve richieste di informazioni e di aiuto direttamente dall'utenza; vaglia e seleziona le chiamate ritenute attendibili ed avvia procedure per mettere in contatto le vittime con le postazioni locali e, successivamente, con gli operatori dei progetti. Il Ministero dell'interno ha poi promosso protocolli d'intesa interistituzionali nell'ambito delle misure di contrasto dell'abuso e dello sfruttamento dei minori, che hanno conosciuto un importante sviluppo e realizzato una serie di eventi formativi e corsi di aggiornamento interni relativi ai reati in danno di minori. Tra le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento delle Forze di polizia operanti nel contrasto della tratta degli esseri umani, va evidenziato il progetto per la «Realizzazione di un *network* e di un intervento formativo comune per funzionari di Polizia, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali sulla lotta alla tratta di esseri umani», il quale progetto è giunto ormai alla sua fase conclusiva, con la redazione di un manuale per la formazione di personale su tutto il territorio nazionale atto a lavorare in questo campo. Tra le iniziative intraprese dal Ministero della solidarietà sociale in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, si sta lavorando ad una ricerca su «Gli interventi di protezione e di reinserimento sociale per i minori vittime di tratte e sfruttamento sessuale», al fine di offrire un contributo tecnico-scientifico alla conoscenza del sistema degli interventi di protezione e reinserimento sociale di bambini, bambine e adolescenti accolti in Italia e seguiti dai servizi territoriali di accoglienza in quanto vittime di tratta e sfruttamento sessuale. La ricerca si pone l'obiettivo di ricostruire un quadro generale delle varie tipologie di intervento attuate in Italia e di offrirne una valutazione centrata sui bisogni e sul punto di vista del minore. I dati ottenuti offriranno indicazioni importanti ai fini delle politiche di accoglienza e protezione e dei programmi di intervento promossi dalle amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali. Inoltre, attraverso la legge n. 285 del 1997, volta a promuovere la realizzazione di interventi concreti di sostegno al mondo dell'infanzia, sono stati avviati una serie di progetti affidati agli enti locali allo scopo di favorire il contrasto di forme di sfruttamento di minori ed è stato avviato un lavoro di valutazione dell'efficacia dei progetti stessi. Un esempio è stato quello citato del progetto realizzato dal Comune di Roma per il Centro di contrasto alla mendicità infantile. Relativamente all'impegno che il Governo intende assumere per l'immediato futuro, si segnala che la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2007 prevede importanti iniziative al fine di realizzare ulteriori interventi volti a realizzare misure di contrasto del fenomeno dello sfruttamento dei minori. Per quanto riguarda, in particolare, lo sfruttamento del lavoro minorile, si prevede la promozione e il monitoraggio delle attività del tavolo tra Governo e parti sociali per il contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile e della dispersione scolastica. Il tavolo di coordinamento tra Governo e parti sociali è stato già ricostituito nello scorso mese di settembre e prossimamente sarà convocato nuovamente per raccogliere i contributi di tutti i soggetti coinvolti, al fine di un aggiornamento degli obiettivi e delle azioni previste nella Carta degli impegni e nel Protocollo di intesa. La ricostituzione di questo tavolo, quindi, è la base per un efficace coordinamento delle azioni da mettere in atto e, in seguito, per una seria verifica della politica di contrasto e una valutazione dell'impatto delle stesse. Con particolare riferimento al fenomeno della mendicità infantile, la direttiva prevede inoltre la predisposizione di azioni positive di garanzia e tutela dei diritti di cittadinanza di bambini e bambine costretti alla pratica dell'accattonaggio, con la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di progetti di formazione specifici rivolti agli operatori sociali. È utile qui ricordare che uno strumento che garantisce un raccordo operativo tra le varie istituzioni che a diverso titolo si occupano del fenomeno dello sfruttamento dei minori è il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, che ha il ruolo di coordinare le attività di prevenzione e contrasto alla pedofilia svolte da diverse amministrazioni dello Stato, raccordandole con le azioni messe in atto dagli organismi privati operanti nel sociale. Nell'ambito di questo osservatorio, è stato altresì istituito un osservatorio con il compito di monitorare l'elaborazione e la gestione coordinata dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali e locali e dagli organismi, anche non istituzionali, operanti a livello europeo e mondiale, ai fini di una più agevole individuazione delle iniziative da concordare in seno al Comitato. In prospettiva, si prevede la futura istituzione di una banca dati in cui vengano sistematicamente raccolte le informazioni attualmente patrimonio dei diversi Dicasteri. Al problema dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, facili vittime di abusi e sfruttamento, è stata riservata una speciale attenzione, sia a livello centrale che periferico. In particolare, il Comitato minori stranieri non accompagnati, che siede presso il Ministero della solidarietà sociale, ha avviato una serie di iniziative volte non solo all'accelerazione dell'*iter* del rimpatrio, laddove possibile (perché non sempre questo è possibile), ma anche relativamente alla definizione di accordi e di progetti con Comuni ed enti locali, volti a monitorare e valutare il fenomeno dei minori e a promuovere azioni di supporto agli enti locali stessi. Da parte del Comitato dei minori è prevista una campagna di comunicazione sul tema dei minori non accompagnati e un convegno, a breve termine, per ragionare insieme agli enti locali su questo fenomeno. Per quanto attiene, invece, ai Rom e ai Sinti che vivono in Italia (le stime parlano di circa 150.000 persone, di cui circa 70-80.000 cittadini italiani), si può prevedere, come è già stato sottolineato, un rilevante incremento, anche derivante dall'ingresso della Romania nell'Unione Europea. Solo un 30 per cento circa di questi gruppi si può considerare ancora nomade; tutti gli altri sono ormai sedentari, in molti casi da decenni, o in via di sedentarizzazione. Al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti e di affrontare anche il tema della sicurezza (rispetto alla quale l'Italia è stata oggetto di rilievi e raccomandazioni da parte degli organismi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa), il Ministero dell'interno, insieme al Ministero della solidarietà sociale, all'ANCI e alle altre amministrazioni, sta valutando l'opportunità di prevedere un disegno di legge organico sulla materia, che tuteli le caratteristiche e le specificità di questi gruppi culturali, consentendone un'effettiva integrazione nella società di accoglienza. Inoltre, il Ministero della solidarietà sociale ha istituito un tavolo sul disagio sociale di queste popolazioni, al quale partecipano le associazioni rappresentative di queste comunità, nonché le associazioni italiane impegnate nella tutela e nel supporto a queste popolazioni, oltre agli enti locali e alle Regioni, per affrontare le questioni relative alle situazioni di marginalità abitativa, devianza e accesso ai servizi sociali. Presso lo stesso Ministero, con la legge finanziaria 2007, è stato istituito un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati che prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e che sarà in parte utilizzato proprio per progetti a favore dell'inserimento sociale dei bambini nomadi in accordo con i Comuni che hanno la più forte incidenza di questo fenomeno. Abbiamo già avuto un primo incontro con i sette Comuni italiani più interessati a questo fenomeno per stabilire insieme in che modo utilizzare questo fondo e come soprattutto articolarlo su tematiche un po' differenti da una parte all'altra in modo da avviare anche proprio delle azioni pilota in questo senso. Nell'ambito inoltre degli accordi vigenti con alcuni Paesi di immigrazione, quali ad esempio il Marocco, si stanno studiando aspetti specifici rispetto alla tutela dei minori e quindi di implementazione degli accordi stessi a favore di una maggiore tutela dei minori stessi. Esiste l'impegno a sviluppare tali accordi con altri Paesi, anche di nuovo ingresso nell'Unione Europea, quali per esempio la Romania. Infine, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui alla legge n. 451 è attualmente impegnato nella predisposizione del Piano di azione 2006-2008 che sarà presentato su proposta dei Ministri della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia. Nella bozza del Piano sono state individuate azioni di sistema e specifiche azioni di settore e una parte particolare è dedicata a tutte le azioni che riguardano la promozione, la protezione e la tutela dei diritti dei minori, articolate in aree tematiche. L'area «discriminazione e soggezione» è specificamente dedicata alle problematiche legate al fenomeno della mendicità infantile. Gli impegni specifici individuati nell'ipotesi di Piano prevedono l'attivazione di politiche finalizzate all'integrazione dei minori di etnia rom, in particolare attraverso un tavolo che riunisca Governo, associazioni rom e associazioni del privato sociale che lavorano con i minori rom, al fine di stilare un piano di azione per l'inclusione sociale dei minori rom con particolare riguardo all'accesso, all'istruzione e ai servizi sanitari; la diffusione di buone pratiche relative a servizi e interventi realizzati al livello locale; la promozione dell'utilizzo di mediatori culturali negli interventi rivolti ai minori rom; la promozione del *curriculum* scolastico, a partire dal nido d'infanzia fino a tutti i gradi di istruzione; l'inserimento di moduli formativi riguardanti le pari opportunità e gli studi di genere volti a promuovere una consapevolezza su tali temi; l'incentivazione di interventi di formazione sulle pari opportunità e gli studi di genere anche in relazione alla variabile culturale per gli insegnanti, gli educatori e tutti gli operatori coinvolti in progetti e interventi per l'infanzia e l'adolescenza; la promozione della cultura tecnico-scientifica tra le ragazze; la promozione di un'attenzione al genere in tutti gli studi e le ricerche sull'infanzia, sia di tipo qualitativo che quantitativo; la promozione di una revisione dei testi scolastici al fine di eliminare le immagini e le rappresentazioni stereotipate del ruolo dei sessi; la promozione nei mezzi di comunicazione di una rappresentazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze non lesiva della loro dignità e dei loro diritti.

Questi sono mirati alla prevenzione e alla lotta all'abuso e allo sfruttamento dei minori, alla prevenzione e alla lotta del traffico di bambini, bambine e adolescenti per motivi di sfruttamento. Sul tema della lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale dei minori la cooperazione italiana ha perseguito una strategia di sostegno a iniziative antitratta, sia attraverso il contributo volontario annuale alle organizzazioni internazionali sia attraverso il finanziamento di progetti mirati. Per questi motivi le mozioni oggi presentate sono mozioni sulle quali il Governo concorda nello spirito e nella sostanza e per le quali si impegna a dare seguito, attraverso iniziative mirate, a progetti che vadano nella direzione di quanto auspicato dalle mozioni stesse.

Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore della mozione presentata dalla senatrice Burani Procaccini, alla quale ho aggiunto anche la mia firma. I problemi esposti in questo documento sono gravissimi e, a mio avviso, non avrebbero avuto bisogno né di commenti né di spiegazioni. La triste realtà di questi bambini, anche piccolissimi, è costantemente sotto gli occhi di tutti. È un fenomeno che purtroppo si registra in tutte le città italiane da Nord a Sud, certamente con maggior evidenza nelle grandi città. Non ci sarebbe bisogno di documenti parlamentari per sapere che lo sfruttamento dei bambini, costretti a vivere al margine dei marciapiedi a chiedere l'elemosina o a vendere un fiore per una monetina, è un problema assolutamente aperto che non può continuare ad essere trascurato. Il voto favorevole di Alleanza Nazionale alla mozione Burani Procaccini serve anche per dire che assistiamo ad un'indifferenza colpevole e generalizzata della gente; tuttavia è certo che il Parlamento non si può permettere alcun atteggiamento di indifferenza e, in questa ottica, riteniamo che il Governo debba determinatamente attivarsi per contrastare in tutti i modi ogni forma di sfruttamento minorile. Ritengo, inoltre, opportuno in questa sede richiamare l'attenzione dei colleghi sul duplice significato di questa mozione: tutelare i minori delle famiglie appartenenti a comunità nomadi ed evitare che essi cadano nelle maglie della peggiore delinquenza e criminalità. Presidente, colleghi senatori, le mozioni in esame toccano una tematica molto cara all'UDEUR, tanto che ho firmato la mozione che vede come prima firmataria la senatrice Serafini e non ho remore nell'esprimere il nostro voto positivo anche per la mozione n. 60 presentata dall'opposizione. Sono convinto, infatti, che la priorità vada sempre data alle azioni intelligenti poste al servizio dei cittadini e soprattutto che queste ci impongano, come classe politica, di superare i contrasti in nome dello sviluppo del Paese. Nello specifico, la tutela dell'infanzia è dovere morale di tutti, prima ancora che impegno politico. In Italia, nonostante esistano leggi idonee, la condizione dei bambini sfruttati rimane tragica: ad un numero sempre più crescente corrisponde un'età sempre più bassa e spesso l'accattonaggio si consuma davanti agli occhi di tutti. Addirittura, a tutt'oggi, il nostro Paese risulta inadempiente rispetto alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. poter sottrarre anche un solo bambino allo sfruttamento e comunque assicurargli protezione, formazione o le più elementari condizioni di igiene è obiettivo con diritto di precedenza. Per questo, a nome del Gruppo Popolari-Udeur, esprimo voto favorevole.

alla mozione che ha come prima firmataria la collega Burani Procaccini. Per aggiungere un fattore di sensibilità, a completamento di quanto ho detto prima, aggiungo un commento ulteriore sulla Carta di Treviso, che avevo citato in chiusura che, come tutti sanno ormai, fu firmata il 5 ottobre 1990 come strumento per tutelare la dignità e l'immagine dei minori, qualora dovessero essere riportati in articoli di stampa. Mi piace ricordare che questa Carta va molto al di là

carta ha come movimento ispiratore la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1989. Un principio espresso in maniera esplicita è: «Il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione». Carta di Treviso, pregando i colleghi di fare mente locale e di immaginare tutti questi princìpi, questi propositi, questi indirizzi, collegati alle immagini, alle allegorie tragiche che sono state fornite dalle testimonianze di tutti i colleghi: «Per le sue necessità» (dice un altro articolo) «di sviluppo psicofisico», il bambino «ha bisogno di particolari cure e assistenza»; pensiamo ai bambini agli angoli delle strade ed ai semafori. «In tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione il maggiore interesse del bambino e perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati»; pensiamo a quei bambini inseriti nel difficile contesto delle rispettive famiglie. Ancora un altro articolo della carta di Treviso dice: «Nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua *privacy* né ad illeciti attentati al suo onore ed alla sua reputazione»; e pensiamo sempre a come questi bambini vengono sfruttati e abbandonati in mezzo alle strade. L'ultima

appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento». Concludo parlando

Quest'ultimo in particolare ha conseguenze gravissime sul futuro dei bambini. Un bambino che resta fuori della scuola è destinato a diventare un adulto che resta fuori dalla società. Signora Sottosegretaria, per far sì che non abbiamo trascorso un pomeriggio di buone intenzioni, la prego di consegnarci, alla chiusura di questo dibattito, un gesto, un segnale, un progetto concreto, per farci capire che siamo capaci di fare un passo in più e che le nostre non sono state soltanto parole, dette con il cuore, dettate dalla solidarietà, ma un impegno concreto a fare finalmente qualcosa.

senatrice Serafini, ma si riconosce, peraltro, anche nel dispositivo descritto dalle altre due mozioni, perché, dalla discussione di oggi e dalla risposta della Sottosegretaria, appare evidente che noi ci troviamo di fronte ad un problema di eccezionale gravità problema di eccezionale gravità e anche di eccezionale novità. Le cose cambiano di anno in anno, vanno sedimentandosi le situazioni più amare, le situazioni che ci colpiscono (ne parlava anche il senatore Valditara), come i bambini portati dalle madri ai semafori, ma ormai la tipologia dei minori di cui dobbiamo occuparci è abbastanza definita e complessa: si tratta di minori stranieri non accompagnati, già grandicelli; si tratta di minorenni vittime della tratta della prostituzione; si tratta di minori stranieri appartenenti a nuclei familiari irregolari, molto problematici, figli di madri sole, spesso provenienti dal mondo della prostituzione; si tratta di minori richiedenti asilo, si tratta di minori segnalati dall'area penale (questo numero sta diventando molto grande). La Sottosegretaria ha risposto, a noi pare in modo positivo, ai due punti finali che si trovano nella mozione della senatrice Serafini.

Ha parlato di una sorta di tavolo di coordinamento delle pratiche migliori. Ciò è molto importante. Io, ad esempio, vengo da una città, Torino, che ha una sorta di primato

Essi vengono rimpatriati e seguiti per sei mesi da associazioni, organi dello Stato italiano o del Comune, da associazioni del Paese d'origine. Si tratta di situazioni molto complesse e costano molto: sei mesi di lavoro sociale e politico. inoltre fatto riferimento a una speciale formazione, promozione e sensibilizzazione non solo dei servizi sociali, che fanno il possibile e l'impossibile, ma anche dei vigili, delle forze di polizia e di quei punti di osservazione e di controllo sociale sul territorio, non allertando i quali poi la madre non la si trova; la si conduce una volta dai vigili o dalla Polizia; la si diffida una volta, ma la seconda volta non la si trova più e, se non la si trova una seconda e una terza volta, non si passa poi alla tutela, all'affido o all'adozione. Esiste una sorta di gioco al rimpiattino, se non si allerta il sistema di vigilanza e controllo anche delle forze di polizia e dei vigili di quartiere, ai quali poi il servizio sociale territoriale e il servizio dei minori si rivolge, ma solo nella misura in cui la segnalazione avviene, è rapida, è puntuale ed è pertinente. Se tutto ciò non accade, il sistema non funziona. a Torino, ad esempio, vi è un servizio di tutela dei minori stranieri che lavora 365 giorni su 365, giorno e notte; 24 ore per 365 giorni. me è capitato più volte di trovare una bambina rom di cinque anni che chiede l'elemosina davanti al «Carrefour» e di telefonare più volte. Vedo che le nostre mozioni parlano di 450 segnalazioni annue. Ciò è impossibile:

più bisognosi di cure, di più certezza della possibilità di ricevere le stesse cure. Il rapporto con il tribunale dev'essere molto puntuale. Crediamo che oggi il Senato abbia svolto un buon lavoro e un alto lavoro; forse non interesserà molto i cronisti, ma finalmente quel senso di pietà e di disagio che coglieva ognuno di noi nelle grandi città del Nord, e molto di più a Roma, ha oggi trovato un momento di riflessione e di proposta adeguata.

finisce qualche volta per uccidere il paziente. Esiste sicuramente una cultura della tolleranza,

Infatti, sicuramente le misure contro la tratta della persona hanno individuato una fattispecie legislativa di rilievo, con pene estremamente importanti;

che crediamo vada rivisto, con realismo, ma anche con senso del dovere. Esistono dei limiti; esiste, ripeto, un senso di responsabilità individuale. Non esiste solamente la responsabilità collettiva, la colpa della società, un qualcosa che non colpisce nessuno. Certo, ogni situazione di degrado va vista in un determinato contesto,

per il reato sulle mutilazioni genitali; non possiamo dare alibi e giustificazioni più di tanto. Per questo, crediamo che su questo aspetto del limite oggettivo, che va posto, e delle responsabilità individuali

perché abbiamo fretta, perché vogliamo andare, ed evitiamo di intervenire in quei casi dove i minori sono al seno o dove non si sa di chi siano, perché in qualche modo ci penserà la società. Ebbene, è un qualcosa che forse non va a nostro merito, ma un limite dovremmo porlo. Pertanto, noi crediamo, onorevole Sottosegretario, che si possa trovare uno spazio per prevedere un reato specifico di impiego di minori nell'accattonaggio, proprio per poter stabilire un limite.

Votiamo invece contro la mozione

difficilmente supportabile oggi nella realtà, ma non aggiungono niente al destino dei bambini. *(Applausi Signor Presidente, innanzitutto volevo ringraziare il Governo per aver rivolto un'attenzione puntuale e particolare a questo fenomeno che,

possiamo cogliere l'invito del Governo ad una valutazione positiva di tutte e tre le mozioni proprio in questo senso, quello cioè di mettere insieme una serie di

lo sfruttamento dei bambini quando avviene ad opera della famiglia (quindi, quando lo Stato deve intervenire con un sostegno e con la prestazione di servizi che accompagnino la famiglia a prendersi la propria responsabilità nei confronti di questi bambini e ad evitare comportamenti illeciti) e quando invece esso avviene ad opera di terzi e quindi dobbiamo intervenire con la repressione massima

perché condividiamo lo stesso punto di vista e riteniamo che sul problema dei diritti negati dell'infanzia non debbano esserci fratture.

ringrazio tutti i colleghi e le colleghe che sono intervenute, nonché la rappresentante del Governo, la sottosegretario

Sono stati ricordati molti dati all'interno di quest'Aula e tutti servono per conoscere e capire quel che avviene, purtroppo, anche sul nostro territorio. L'Organizzazione internazionale del lavoro, per esempio, stima che nel mondo ci siano più di 250 milioni di bambini sottoposti allo sfruttamento lavorativo.

Di questi 250 milioni, pare che più della metà abbia un'età compresa tra i 5 e i 15 anni, come ricordava anche la collega Serafini. Di fatto, però, non stiamo parlando solo dello sfruttamento lavorativo, che sarebbe già una sorta di obbrobrio, di problema inaccettabile, ma di qualcosa che colpisce,

che tutti noi oggi diciamo di non accettare. Per questo ci assumiamo degli impegni e delle responsabilità.

Quale fotografia emerge? Emergono sostanzialmente dei bambini, delle bambine, degli adolescenti, da 0 (perché in alcuni casi si tratta di bambini di pochissimi mesi tenuti tra le braccia

di carattere sessuale. Ho sentito parlare la Sottosegretario e alcuni dei colleghi di tratta degli esseri umani, che sicuramente rientra anche all'interno di questa fattispecie, soprattutto di persone cui viene tolta la possibilità di essere soggetto umano, sottoposto allo scherno dell'opinione pubblica; di persone prive della possibilità

l'Italia, attraverso queste mozioni, si assuma oggi qualche responsabilità in più. Siamo consapevoli che non riusciremo a debellare questo problema e questo fenomeno, però sappiamo che le nostre leggi sono delle buone leggi;

che ha istituito il primo vero fondo per l'infanzia e l'adolescenza, proprio per porre attenzione alle condizioni di normalità, ma anche a queste condizioni di drammatica non normalità per i bambini e gli adolescenti.

del *welfare* e della solidarietà, c'è bisogno sicuramente del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione

facciamo fatica a individuare le soluzioni più efficaci. Ci sembra un problema drammatico ma, onestamente, sia a livello italiano che europeo, stiamo facendo fatica a individuare dei percorsi di accoglienza e di inclusione sociale per molti di questi bambini.

deve essere rivolto un di più di attenzione, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, e, fatto non secondario, la disponibilità all'ascolto delle opinioni del bambino. Veniva ricordato da alcune colleghe che, prima che venisse emessa la sentenza della Cassazione succitata,

in questa sede il nostro forte contrasto ad ogni forma di violenza esercitata sui bambini e ad ogni forma di accattonaggio e di sfruttamento minorile. Pertanto, esprimiamo, con convinzione, senatrice Serafini, e alle altre mozioni per dire no a queste disumane forme di violenza verso i bambini e gli adolescenti.

oltre che dell'attacco, anche del ferimento di un nostro soldato presente in Afghanistan, io sono a chiedere a lei d'intervenire presso il Governo perché il ministro Parisi possa riferire pure su questo episodio evidentemente molto grave,

Signor Presidente, preferisco leggere una nota perché il tema è abbastanza complesso e di natura tecnica. questo ci può aiutare a comprendere meglio il problema che si sta creando in merito agli ufficiali della Marina militare, ma anche alle altre Forze armate. La Marina militare arruola ufficiali in ferma prefissata con il concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002.

Tali ufficiali, in servizio da ottobre 2003, sono da considerarsi precari storici poiché, come gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, sono in servizio da almeno tre anni, o conseguiranno tale requisito grazie ad un provvedimento relativo al 2006. Attualmente, con tale requisito sono in servizio circa 200 ufficiali in ferma prefissata dei primi quattro corsi. La legge finanziaria del 2007, proprio nell'affrontare il problema dei precari storici con contratto a termine di tre o più anni, prende in esame anche il personale

hanno arruolato ufficiali in ferma prefissata per mezzo di tale decreto. L'articolo 1, del comma 519 della legge n. 296 del 2006

Il comma 519 non cita esclusivamente gli allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, ma si riferisce a tutti gli ufficiali in ferma prefissata enunciati nell'articolo 23, comma 1 del sopra citato decreto. L'ipotesi di escludere dalla stabilizzazione gli allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina Militare e delle altre Forze armate costituirebbe una evidente illegittimità costituzionale del comma 519, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra ufficiali delle Forze armate. Gentili colleghe, vi prego di farmi parlare.

Al fine di attuare la professionalizzazione delle Forze armate, sono state istituite diverse forme di volontari, tra essi gli ufficiali in ferma prefissata. Questi sono dei dipendenti del Ministero della difesa che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, una tipologia di rapporto da distinguersi da quelle forme di servizio prolungato esistenti nelle Forze armate. l'ufficiale in ferma prefissata è iscritto all'INPDAP, fin dal primo anno ha diritto a licenza ordinaria, percepisce la tredicesima e il trattamento di fine servizio alla fine del contratto a tempo determinato. Da ciò si può facilmente dedurre che sono dei dipendenti pubblici a termine come gli altri precari delle amministrazioni militari e civili, pertanto, a tali ufficiali deve essere assicurato lo stesso trattamento giuridico degli altri lavoratori pubblici precari. Proprio per tale motivo, l'Arma dei carabinieri attua il principio della stabilizzazione enunciato dal comma 519 al fine di garantire un futuro ai propri ufficiali precari. la Marina militare ha arruolato ufficiali in ferma prefissata. Tali ufficiali precari, che hanno più di tre anni di servizio, hanno lo stesso *status* giuridico e un trattamento economico, matricolare e previdenziale uguale agli altri precari pubblici. Nel periodo in cui è stato istituito il fondo, di cui al comma 96, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non esisteva ancora un precariato storico con le stellette; la finanziaria nel 2005 ancora non aveva istituito il diritto alla stabilizzazione per i precari con contratto a tempo determinato da almeno tre anni.

con oltre tre anni di servizio, anche in virtù delle recenti sentenze della Corte di giustizia europea. Un altro elemento comune, sia all'Arma dei carabinieri, sia alla Marina militare è che gli ufficiali in ferma prefissata dei primi corsi hanno più di tre anni di servizio o maturano tale requisito per effetto di proroghe intervenute prima del 31 dicembre 2007. Un'esclusione alla stabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata della Marina militare determinerebbe quindi una disparità di trattamento, poiché sono entrambi nella stessa condizione giuridica avendo entrambi un contratto a tempo determinato per più di tre anni. Gli ufficiali in ferma prefissata della Marina militare con due anni e sei mesi di servizio sono quelli appartenenti al V corso, che sono stati congedati il 5 marzo 2007, mentre i primi quattro corsi hanno oltre i tre anni di servizio o conseguiranno tale requisito in virtù dei contratti stipulati prima del 29 settembre 2006. Tra questi ufficiali vi sono dei giovani, ma non troppo, che dopo tre anni hanno acquisito delle competenze tecnico-professionali e sono stati parte attiva dell'amministrazione. Il compito dell'ufficiale a ferma prefissata non è stato solamente quello di sostituire l'ufficiale di complemento, infatti sottotenenti di vascello dei ruoli normali hanno ricoperto incarichi svolti da ufficiali in servizio permanente. Non bisogna dimenticare che l'Arma dei carabinieri ha impiegato degli ufficiali in ferma prefissata nei servizi ricoperti prima dagli ufficiali di complemento. Il concorso in ferma prefissata prevedeva, quale limite d'età, quello dei 38 anni, pertanto la Marina militare non voleva assumere dei giovani ragazzi senza esperienza, bensì soggetti con elevato bagaglio professionale, costituito da un alto titolo di studio e da una provata esperienza lavorativa. Gli ufficiali in ferma prefissata della Marina militare non hanno avuto la possibilità di transitare nel servizio permanente, visto che da quando è stato arruolato il primo corso di allievi ufficiali in ferma prefissata sono stati banditi concorsi per ruoli speciali con numero di posti palesemente esigui e senza riserve. Solo il Genio navale e i sanitari hanno bandito, per pochi posti, dei concorsi per il ruolo normale per il servizio permanente. Proprio in virtù della riduzione dei finanziamenti, è giusto sottolineare che nessuna azienda che opera una riduzione di spesa licenzierebbe personale qualificato per poi assumerne altro con i relativi costi per il reclutamento e l'addestramento. Ci troviamo chiaramente di fronte ad un *turnover*, signor Presidente, colleghi, perché è impensabile poter parlare di ulteriore aggravio di spesa nel momento in cui ormai siamo al V corso e puntualmente si ritengono necessari ed indispensabili questi soggetti e non si capisce il motivo per il quale si stia creando un processo assurdo a produrre solo e soltanto precari, dove si formano per tre anni, si investe su queste persone e, nel momento in cui possono operare con la capacità e con la titolarità d'azione, puntualmente vengono mandati a casa per assumerne altrettanti, tenerli altri tre anni, continuare formarli per poi mandarli a casa e così via, siamo già al quinto corso e credo che dovremmo mettere un fermo a tutto questo.

solamente per l'Arma dei carabinieri, non per i marinai, che vengono considerati del ufficiali di serie B, senza diritto di stabilizzazione. Se poi la finanziaria 2007 non si applica al personale militare, sarebbe interessante sapere perché agli ufficiali del V corso non è stato riconosciuto il diritto dell'anno di rafferma, cosa che avrebbe consentito loro di maturare il requisito dei tre anni di servizio previsto dal comma 519 e pertanto, in data 5 marzo 2007, sono stati congedati dopo aver terminato la ferma dei 30 mesi. In conclusione, si ritiene che, essendo stato sospeso il servizio militare obbligatorio, il reclutamento ed il regime dei contratti degli ufficiali in ferma prefissata debba essere adeguato alle regole che il mercato del lavoro prevede per coloro che siano stati assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato e è inoltre obbligo che tutte le amministrazioni statali debbano rispettare le normative che regolano e sanzionano un utilizzo abusivo di successione e di contratti di lavoro a tempo determinato. Con questo voglio solamente sottolineare come andremmo a punire, laddove si volessero determinare, in soggetti privati, un concorso continuo con contratti a tempo determinato, paradossalmente l'amministrazione statale sta facendo un'azione che produrrà, come sta producendo, situazioni che vanno sicuramente sanate. Ecco il motivo per il quale mi auguro che la mozione venga accolta e che il Governo trovi una soluzione adeguata per queste persone, per questi professionisti che hanno dato e si sono formati grazie anche ad un supporto corretto dell'amministrazione, sia della Marina militare, ma anche delle altre Forze armate.

Ricordo che il problema del precariato degli ufficiali non è nuovo; nel recente passato ha investito ben un ventennio della nostra storia. Ci sono volute numerose leggi per arrivare a quel ruolo ad esaurimento che ha sanato tutto il contenzioso degli ufficiali di complemento, prima trattenuti, poi raffermati. Questo processo ha creato, tra l'altro, malumori tra ufficiali dei ruoli normali e delle accademie e quelli del ruolo ad esaurimento per le diverse attribuzioni nel grado e per la differenza di trattamento riguardo ai requisiti per la progressione delle carriere, innescando rivendicazioni sia da una parte che dall'altra. È accaduto che ufficiali dei ruoli normali sono stati scavalcati da ufficiali del ruolo ad esaurimento, perché i primi dovevano sostenere prove e attribuzioni specifiche che ai secondi non erano richieste. Dall'altra parte, ufficiali di provata esperienza e di notevole competenza non potevano assumere incarichi di responsabilità perché l'appartenenza al ruolo ad esaurimento non lo consentiva. Memori di questa esperienza, che succintamente ho richiamato, evitiamo di ricadere negli stessi errori. Con il passaggio al sistema interamente professionale, la leva obbligatoria è stata sospesa, quindi gli ufficiali di complemento, cioè il loro equivalente rappresentato dagli attuali arruolamenti in ferma prefissata, transitano ad un rapporto di impiego a tempo indeterminato. In questa legislatura il Governo aveva già assunto un impegno riguardo agli ufficiali dei carabinieri: impegno ad assumere utili iniziative affinché gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, la cui ferma doveva concludersi definitivamente negli anni 2006 e 2007, potessero essere raffermati a domanda per un ulteriore periodo. In sede di approvazione del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, dove si prevedeva il prolungamento fino al 31 dicembre 2006 del trattenimento in servizio di 1.316 agenti ausiliari della Polizia di Stato che avevano frequentato il sessantatreesimo il Governo onorò l'impegno preso e gli ufficiali dei carabinieri in ferma prefissata furono trattenuti fino al 31 dicembre 2006. Ma anche nella precedente legislatura questo problema era già emerso. Ricordo che nel corso del dibattito relativo all'Atto Senato n. di conversione del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, riguardante la stabilizzazione degli agenti ausiliari frequentatori del sessantunesimo, sessantaduesimo corso, fu approvato al Senato un emendamento di cui ero primo firmatario. riguardava, appunto, proprio la possibilità di bandire concorsi per l'ammissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri in maniera adeguata rispetto al numero in servizio, poiché, su circa 500 ufficiali in ferma prefissata, si prevedeva il passaggio in servizio permanente per solo cinque di loro. L'altro ramo del Parlamento non ratificò l'emendamento perché il Governo, che al Senato si era rimesso al volere dell'Assemblea, inspiegabilmente alla Camera si oppose. Un dato politico era emerso, quindi, già nella precedente legislatura; vi erano e vi sono forme di precariato anche nelle Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. Il precariato è entrato, quindi, prepotentemente prima nel programma dell'Unione, poi nell'agenda di Governo. È infatti grazie alla legge finanziaria, la quale prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione a tempo determinato, che fosse in servizio al 31 dicembre 2006, che abbia maturato almeno tre anni di servizio o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, che noi della noi della maggioranza, oggi, insieme anche all'opposizione, abbiamo ritenuto di presentare la mozione a firma Nieddu e altri riguardante tutti gli ufficiali in ferma prefissata di tutte le armi, e quella a firma del senatore Tofani, che mi ha preceduto poc'anzi, per gli ufficiali della Marina militare, oggi in discussione. La mozione da noi presentata, oltre a chiedere di dare continuità al rapporto di servizio degli ufficiali in ferma prefissata per consentir loro di maturare i tre anni di servizio, condizione necessaria per avere diritto alla stabilizzazione, propone al Governo di assumere iniziative, anche di carattere legislativo, con l'obiettivo di collocare presso altre amministrazioni dello Stato, come, per esempio, la Protezione civile (dove sappiamo c'è l'esigenza di personale del quadro intermedio), previo consenso degli interessati, personale militare più anziano, eventualmente in esubero, allo scopo di liberare posti in organico da far ricoprire agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate, creando così le condizioni per un'eventuale trasformazione del rapporto di servizio dei predetti da tempo determinato a tempo indeterminato. Ciò consentirebbe di continuare a impiegare questi giovani ufficiali non disperdendo un patrimonio speso per formarli, dando il tempo necessario al Governo per mettere in atto le azioni utili a sanare definitivamente la situazione. Infatti, se risponde al vero che sono 1.800 gli ufficiali che si trovano in questa condizione di contratti di servizio a tempo determinato, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è anche vero che il numero degli ufficiali (circa 25.834) risulta oggi squilibrato rispetto al modello di difesa esistente ed ancor più rispetto a quello in corso di definizione; 25.834 ufficiali su 193.000 unità totali di Esercito, Marina e Aeronautica significa meno di un ufficiale ogni otto unità circa. Dunque il problema è quello di ringiovanire i ruoli degli ufficiali e non solo di dilatarne il numero. Il problema va visto anche sotto un altro aspetto. Gli ufficiali in ferma prefissata sono soggetti ad un contratto della durata di trenta mesi, che non consente, quindi, in prima istanza il diritto alla stabilizzazione, cui si accede dopo trentasei mesi. Dunque, 1'amministrazione può dare continuità al rapporto di servizio dei predetti ufficiali concedendo loro un'ulteriore rafferma di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 8 maggio 2001, n. 215. Va quindi valutata per i militari di cui stiamo parlando la possibilità di essere raffermati per ulteriori dodici mesi allo scopo di maturare il diritto alla stabilizzazione. Infatti, sarebbe paradossale che una norma costruita per tutelare il personale si ribaltasse nel suo opposto; non credo sia questo lo spirito della legge. Certo, ci saranno delle valutazioni di merito che il Governo in proposito dovrà fare. Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, la previsione normativa relativa alla stabilizzazione è esplicitamente richiamata nelle norme citate. Peraltro - mi avvio alla conclusione - occorre tenere conto che è anche allo studio una riorganizzazione del modello di difesa, cui facevo cenno, e quindi degli organici di Esercito, Marina e Aeronautica. Questo, signor Presidente, colleghi e colleghe, è il contesto nel quale poniamo l'esigenza di questo di indirizzo al Governo. Ci rendiamo conto che il conseguimento della soluzione sta dentro un'articolata pluralità di azioni, che consentano il passaggio in servizio permanente dei giovani ufficiali, e allo stesso tempo il mantenimento di un accettabile equilibrio tra il ruolo degli ufficiali, quello dei sottufficiali e quello della truppa. È per queste ragioni che ho consegnato alla Presidenza la riformulazione del dispositivo della mozione che avevo depositato per l'esame di questa onorevole

Con le mozioni in discussione i senatori proponenti affrontano la complessa tematica riguardante gli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate, in particolare quelli della Marina militare, e chiedono con i relativi atti di indirizzo un impegno del Governo ad assumere urgenti iniziative volte a prevedere che il predetto personale possa transitare nel servizio permanente effettivo, a dare continuità al rapporto di servizio degli ufficiali in ferma prefissata, concedendo loro un'ulteriore rafferma di dodici mesi e ad assumere iniziative anche di carattere legislativo con l'obiettivo di collocare presso le amministrazioni dello Stato, previo consenso degli interessati, personale militare più anziano eventualmente in esubero allo scopo di liberare posti in organico da far ricoprire agli ufficiali in ferma prefissata nelle Forze armate. In attuazione a quanto disposto dal decreto-legislativo n. 215 del 2001, ogni Forza armata può reclutare ufficiali in ferma prefissata della durata di due anni e sei mesi prorogabili di un ulteriore anno, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate che necessitano della presenza di un'aliquota di personale che, per età e condizioni fisiche, sia idonea ad assolvere i compiti strettamente operativi. Si evidenzia in questo modo che il ricorso agli AUFP ha come precipua finalità quella di garantire alle Forze armate, per un predeterminato e limitato periodo di tempo, l'utilizzo di specifiche professionalità atte a soddisfare rapidamente particolari esigenze operative. La temporaneità del rapporto d'impiego che lega il militare all'amministrazione è quindi funzionale a precise esigenze istituzionali ed è stata prevista dal legislatore anche al fine di evitare che un eccessivo prolungamento della ferma possa ingenerare negli interessati ingiustificate aspettative di una stabilizzazione del rapporto stesso. Occorre osservare al riguardo che il carattere di temporaneità, che caratterizza questo rapporto d'impiego, è ben noto agli interessati, che prendono parte alle procedure concorsuali dopo aver preso conoscenza e accettato le modalità e le condizioni previste dai relativi bandi. Peraltro, in un tale quadro, va fatto rilevare che un'eventuale immissione *sic et simpliciter* nel servizio permanente di tale fattispecie di personale avrebbe sicure ripercussioni sulle dinamiche dei reclutamenti ordinari, in quanto inciderebbe sulle progressioni di carriera nei vari ruoli nonché sulle connesse pianificazioni di impiego del personale ufficiale di Forza armata. Ciò posto, i commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 recano disposizioni per la stabilizzazione di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazione in servizio a tempo determinato, purché in possesso di determinati requisiti. In particolare, il primo periodo del citato comma 519, prevede in generale un programma di stabilizzazione di lavoratori precari che siano in servizio da almeno tre anni o che conseguano tale requisito per effetto di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, ovvero che nei cinque anni antecedenti al 1° gennaio 2007 siano stati in servizio per almeno un triennio. Il successivo terzo periodo di tale comma, inoltre, dispone che le amministrazioni continuino ad avvalersi del personale in argomento e in maniera prioritaria del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo dell'8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni - in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Il programma di stabilizzazione volto al comune precariato storico prodottosi nel tempo in ambito pubblico è finanziato con una quota delle risorse per il fondo per le assunzioni nel pubblico impiego. Al riguardo, al personale delle Forze armate non si applicano le disposizioni di carattere generale riguardanti le assunzioni nel pubblico impiego in quanto tale materia è segnatamente disciplinata dalla normativa di settore che ha già determinato al 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna categoria di personale e che, nel periodo transitorio, demanda annualmente ad uno specifico decreto di concerto (Difesa, Economia, Funzione pubblica), la determinazione delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale dell'esercito della Marina e dell'Aeronautica nel rispetto dell'entità complessiva di 190.000 unità e compatibilmente con l'evoluzione degli oneri autorizzati. Per tale ragione, le Forze armate sono state escluse dal blocco delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2005 e conseguentemente dall'utilizzo del fondo per le assunzioni in deroga. Relativamente agli ufficiali in ferma prefissata, si sottolinea, come già evidenziato, che il loro reclutamento ha come finalità quella di garantire alle Forze armate, per un periodo predeterminato e limitato di tempo, l'utilizzo di professionalità tecniche che, per età e condizioni fisiche, sono idonee a fronteggiare rapidamente particolari esigenze operative. Il carattere temporaneo costituisce quindi il connotato essenziale di tale rapporto. Pertanto, la priorità alla stabilizzazione del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 215, prevista dal comma 519 della legge finanziaria 2007, è da intendersi riferita unicamente agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri e della Guarda di finanza. Con riferimento poi agli ufficiali ausiliari in ferma prefissata appartenenti al V corso di cui si fa cenno nella mozione, si fa presente che la Marina militare non si è avvalsa della facoltà prevista dall'attuale legislazione di attivare le procedure per la conferma per un ulteriore anno a seguito di tali tagli, infatti infatti tutte le Forze armate, compresa la Marina, hanno dovuto rivedere in chiave riduttiva i volumi di reclutamento previsti per il 2007. A ciò si deve aggiungere un elemento di criticità di non minore importanza costituito dalla esiguità delle risorse finanziarie messe a disposizione, dei mezzi e sistemi atti all'assolvimento dei compiti istituzionali di difesa nazionale e di mantenimento della pace nell'ambito delle varie missioni internazionali. Concludendo, quindi, Concludendo, quindi, il Governo esprime parere favorevole alla riformulazione della mozione del senatore Nieddu e parere negativo sulla mozione del senatore Tofani.

Signor Presidente, colleghi senatori, dichiaro, a nome del Gruppo che rappresento, il voto favorevole alla mozione n. 80 del centro-sinistra e chiedo di consegnare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.

esattamente che vi rientrano anche le Forze armate, in modo particolare ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guarda di finanza. Pertanto, ancora una volta emerge la volontà di discriminare alcuni militari che si trovano in condizioni tali da poter trovare una soluzione proprio per quella norma che nella finanziaria è stata approvata, cioè il comma 519, che prevede la stabilizzazione a domanda di quei soggetti che hanno dei requisiti, e cioè almeno tre anni di anzianità. Ne prendo atto anzianità. Ne prendo atto con rammarico e interpreto il sentimento di tutti questi militari che si sentono esclusi e danneggiati

evasivo, soprattutto perché entra in un merito in cui difficilmente potremo trovare riscontro di competenze in un'Aula parlamentare. Mi sembra che tale dispositivo voglia rappresentare solamente un elemento sia pure di attenzione, ma senz'altro non di certezza per i soggetti per i quali oggi stiamo dibattendo e discutendo. Sono soddisfatto che Alleanza Nazionale e il sottoscritto abbiano posto all'attenzione un problema così importante, che purtroppo veniva marginalizzato se non addirittura celato. Mi auguro che vi possa essere maggiore attenzione da parte del Governo. Per quanto concerne il voto, spero che i colleghi in Aula vogliano votare anche la mozione che mi vede quale primo firmatario, anche perché nel dispositivo della mozione, signor sottosegretario Verzaschi, si afferma: «Impegna il Governo ad assumere urgenti iniziative volte a prevedere che il predetto personale possa transitare nel servizio permanente effettivo, anche per restituire legalità, serenità e chiarezza alle centinaia di giovani ufficiali in ferma prefissata della Marina militare.»

perché essa non rappresenta concretamente un percorso che possa dare garanzie. Mi auguro che i colleghi vogliano, secondo coscienza, valutare il voto della mozione che mi vede quale primo firmatario sperando di avere consenso.

allora è molto seria e di conseguenza deve essere documentato chi in quest'Aula, di fronte ad un Paese impegnato su teatri di guerra, e non di pace, come l'Afghanistan, vuole fornire mezzi, risorse,

chiesta: avevo chiesto io il voto elettronico e se lei guarda tra coloro che hanno votato vedrà che non ho potuto esprimere il mio voto perché la scheda non mi era ancora arrivata. Quindi, mi pare sia questa la dimostrazione...

Signor Presidente, lei ha detto cose tutto sommato condivisibili, ma c'è un piccolo particolare: faccio riferimento alle modalità di votazione previste dal nostro Regolamento

In questo caso, la richiesta di votazione elettronica non è stata avanzata da un qualunque senatore, ma dal Presidente di un Gruppo parlamentare che si presume abbia la rappresentanza del Gruppo medesimo, come è prassi costante nei lavori parlamentari in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento.

che questa costituisca un precedente. Molte volte è successo che, per motivi vari, ci sia stata una divaricazione di iniziative; ad esempio, io son di quelli che non han capito se dovevano votare o no perché sono arrivati all'ultimo istante. Credo debba prevalere sempre

la mozione è respinta.

Grazie,